prevedeva la piena parità tra uomini e donne in materia di lavoro; tale legge ha fatto sì che il dettato costituzionale, e in particolare gli articoli 3 e 37, fosse finalmente applicato in ambito lavorativo. Sua ancora è la legge n. 833 del 1978 sul Servizio sanitario nazionale: da Ministra della sanità, dopo essere stata per due anni Ministra del lavoro, lavoro, realizzò e unificò il Servizio sanitario nazionale. Non è di poco conto ricordare questo importante quarantesimo anniversario, il Paese ancora oggi vede un sessismo strisciante nei confronti di donne impegnate in politica. Vi è, tuttavia, un'esperienza che desidero ricordare più di tutte,

L'austera, l'onesta figura di Tina Anselmi non a caso è stata indicata per rappresentare, con la sua indispensabile autorevolezza e con il suo grande senso dello Stato, la Commissione volta a restituire dignità a istituzioni infiltrate e calpestate.

Solo frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci viene delegato dal popolo, possa essere ridotto a una mera appartenenza. La P2 si è impadronita delle istituzioni, ha fatto il colpo di Stato strisciante. Per più di dieci anni i servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto». noi ricordiamo Tina Anselmi per dire oggi, pur essendo lei in vita anche se gravemente malata, che la verità possono cercarla davvero solo coloro che riescono a sopportarne le conseguenze. Ce ne rendiamo conto ogni giorno e oltre ogni pregiudizio non dobbiamo stancarci di lottare per cercare verità e sostenere quella democrazia per cui lei ha lavorato così profondamente e in modo così convinto, così a rischio e così consapevole. Grazie Tina. La Presidenza si associa a questo apprezzamento, ma voglio dire che spero Tina Anselmi ci stia seguendo. Le mandiamo tutti insieme un grande abbraccio.

Presidente, preliminarmente alla seduta che sta iniziando si è svolta una riunione informale della Commissione agricoltura che ritengo molto utile nell'auspicio e certamente anche nel predicato. L'obiettivo era quello di giungere a una sintesi tra tanti emendamenti, a una proposta che, modificando questo provvedimento legislativo e integrandolo con il contenuto degli emendamenti, lo rendesse meritevole del sostegno

che, se fosse valutato favorevolmente da parte del Governo, ci porterebbe a ritirare tutti gli emendamenti presentati a firma del sottoscritto o di altri senatori del Gruppo Lega Nord. Questo per una ragione molto semplice: è un provvedimento importante, che deve essere agevolato nel suo cammino di attuazione, ma che non può trascurare le difficoltà cui può andare incontro il mondo dell'agricoltura onesto, quello che lavora già seguendo le regole.

un testo 2, siamo disposti anche a modulare diversamente l'emendamento, ma questa è la proposta che rinnovo al Governo: considerare l'emendamento 8.0.205, su cui credo anche i senatori delle Autonomie avranno qualcosa da dire.

non prevista dal nostro Regolamento, che è stata a lungo dibattuta anche quando trattammo della riforma costituzionale. In quella occasione, il Presidente riconobbe, alla fine del dibattito, che bisognava procedere articolo per articolo.

per motivi che a qualcuno possono sembrare arcani, ma che per gli addetti ai lavori sono molto chiari (la maggioranza teme di non avere i numeri all'interno di quella Giunta), non viene mai convocata. Abbiamo decine di quesiti per i quali abbiamo chiesto la convocazione della Giunta per il Regolamento e puntualmente questa nostra richiesta è stata disattesa. Più volte ho detto, anche in quest'Assemblea, che la creazione di precedenti, nella volontà della maggioranza, oggi come oggi sposta poco, perché non ci saranno Senati susseguenti, almeno nella volontà di questa maggioranza; poi vedremo se, nella volontà del popolo italiano, ci sarà ancora un Senato come questo oppure qualcosa di diverso (qualche brutta fotocopia).

l'illustrazione cumulativa degli emendamenti, anche perché, nell'articolazione dei disegni di legge, molto spesso alcuni emendamenti di articoli successivi dipendono, nel contenuto e quindi nella sostanza (sempre che si voglia andare alla sostanza dei provvedimenti), dall'esito delle votazioni degli articoli precedenti.

parere conforme a quello della relatrice. L'articolo 1 presenta la fattispecie del reato, tema sul quale si è trovato un punto di sintesi, anche con la Commissione giustizia. Pertanto riteniamo sia importante mantenere tale elemento di equilibrio.

dichiarazione di voto.

ciò di cui si parla deve essere vicino e conseguenziale alle scelte fatte sugli articoli precedenti. Ciò mi sembra doveroso per la serietà dei lavori parlamentari, altrimenti diciamo chiaramente che si tratta di votificio

prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale».

**Il Senato approva**.

Signor Presidente, colleghi senatori, questa Assemblea oggi...

a farlo con celerità per consentire al senatore Stefano di svolgere il suo intervento.

E lo fa approvando un provvedimento che pone le basi ed offre più puntuali e specifici strumenti per combattere il caporalato in agricoltura. a questa pagina ha contribuito - lo voglio riconoscere - la responsabilità e l'approccio della relatrice Gatti, che ci ha consentito

perché ad essere sfruttata da questo fenomeno non è solo la manodopera dell'uomo, che non è mai merce, ma l'intera persona, che viene indebolita e stritolata dalle necessità, dalla povertà, dal bisogno e infine consunta dalla fatica stremante. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è quindi, a mio avviso, un buon punto di partenza. Personalmente, proprio un anno fa, quando nella cronaca si rincorrevano e assommavano le morti di donne e uomini caduti vittime del caporalato, ho fatto mia l'idea di istituire...

Senatore Airola, faccia il bravo. ho fatto mia l'idea di istituire una Commissione d'inchiesta su questo fenomeno. Avevo individuato nella Commissione d'inchiesta uno strumento utile a scandagliare la mutazione genetica che da tempo è in corso e che riguarda le diverse forme di sfruttamento dei lavoratori. Queste forme di schiavitù, infatti, non si registrano solo nei campi. Esistono vere e proprie degenerazioni nel settore dell'edilizia, dei trasporti, dei *call center*, fino ad arrivare a modelli più complessi, come possono essere le cooperative spurie. Ho presentato anche un disegno di legge, che è quello associato al presente, dal quale sono stati presi alcuni spunti che sono andati ad arricchire il testo del Governo che è stato preso a riferimento in Commissione. Abbiamo cercato - ed ho cercato - di contribuire ulteriormente alla miglior riuscita di questo provvedimento, facendomi ulteriormente promotore dell'iniziativa, positivamente accolta dai colleghi della Commissione e dal presidente Formigoni, di proiettare il docu-film «Santi Caporali», girato e prodotto da un giovane regista salentino, Giuseppe Pezzulla. Le immagini toccanti, girate, per ragioni di sicurezza, con un cellulare nel ghetto di Rignano Garganico, ci hanno raccontato quello che accade in quella terra di nessuno: dai giovani africani che vanno a lavorare nei campi ai giovani pugliesi che cercano di alleviare il peso di questo sfruttamento preparando un pasto caldo, distribuendo caramelle e matite ai bambini, insegnando in alcuni casi a leggere e scrivere e aggiustando quelle benedette biciclette. Abbiamo avuto anche l'onore di ascoltare il commosso silenzio di un emozionatissimo giovane, Gora Seck: un giovane sudanese che da anni lavora sotto caporale e che è uno dei protagonisti che si racconta nella pellicola. Non nascondo di nutrire una particolare sensibilità nei confronti di questo dramma, con il quale, prima come cittadino pugliese, poi poi come assessore all'agricoltura e oggi come senatore della Repubblica impegnato in Commissione, mi sono dovuto più volte misurare e che finalmente abbiamo avuto la possibilità ed il coraggio di cominciare ad aggredire in modo sistematico ed efficace. Riconoscendo l'importante lavoro della relatrice, mi ripeto, sono altrettanto consapevole che oggi si è ad un punto di partenza e non di arrivo, ma da qualche parte bisognava pur cominciare. Diciamo quindi che questo, per me, è un momento di grande responsabilità, di corresponsabilità tra Governo e Parlamento del quale quest'Aula deve essere orgogliosa. È per questo motivo che dichiaro il voto favorevole al provvedimento del nostro Gruppo.

Presidente, sarò brevissimo, dopo dieci anni arriva un provvedimento importante e determinante, anche se con molto ritardo perché questa forma di caporalato esisteva già quando i lavoratori ma negli ultimi anni, come sapete, in seguito all'immigrazione, ormai è un fenomeno al 90 per cento non italiano che vede situazioni di degrado incredibili. 400.000 i lavoratori più o meno utilizzati e 100.000 quelli ridotti a livello di schiavitù senza il minimo dei servizi possibili, che riscuotono paghe da fame e che subiscono estorsioni anche per un panino e una bottiglia di acqua minerale. Dunque ben venga questo provvedimento.

Non è possibile: questo significa metterlo in condizioni di subalternità. Bisogna creare un unico organismo di controllo per far sì che l'operatore onesto e corretto sia sereno e tranquillo nell'esercizio della sua attività. Questo dovrebbe essere il minimo. Dovremmo poi cercare di

cioè, in una parola, non possiamo non immaginare che il piccolo produttore agricolo, che ha due o tre ettari, a certi costi non potrà raccogliere. Si dice che non deve pagare? No, deve pagare, ma andiamogli incontro. Io mi rendo conto della difficoltà ma l'operatore agricolo onesto e il piccolo operatore devono essere aiutati con la diminuzione della tassazione o con aiuti. Le difficoltà finanziarie ci sono tutte ma vanno affrontate altrimenti il piccolo operatore lascerà il prodotto lì, con il danno che ne deriva il grande subirà danni inauditi, questo è il dato reale. Una politica vera nei confronti degli operatori onesti in agricoltura non c'è ed è questo l'invito che faccio al Governo.

se qualcosa andrebbe modificato nei Regolamenti parlamentari è proprio il fatto che se il Governo si impegna con gli ordini del giorno poi dovrebbe impegnarsi a rispettarli altrimenti se ne perde il significato. Questa nuova norma sul caporalato è da molto tempo attesa è certamente un'apripista importante ma non credo che sarà conclusiva ed esaustiva della questione proprio perché inquadrare realmente il caporalato, in tutte le sue tristi dinamiche, è cosa assai difficile.

Ne abbiamo discusso anche in Commissione: definiamo delle regole per le quali si dovrebbe avere un prodotto in agricoltura che non è stato conseguito utilizzando modalità scorrette e offensive della dignità umana come quelle del caporalato.

Dal mondo dell'agricoltura sono state avanzate delle proposte emendative che tengono conto della differenza che c'è nel fare agricoltura nel nostro Paese.

poco meditata nella fase conclusiva, si vada a rendere la vita difficile a chi le regole già rispetta. Ed è cosa tipica del nostro Paese: si fa una legge

settimana scorsa, il Ministro dall'agricoltura ha fatto il suo comunicato stampa, dopo che in una seduta notturna in Commissione erano stati respinti tutti gli emendamenti, sia quelli presentati quelli presentati dai Gruppi di opposizione sia qualcuno presentato da Gruppi di maggioranza, al solo scopo di poter dichiarare, prima della pausa estiva, che il Governo ha ha fatto proprio un provvedimento che vuole risolvere il problema del caporalato. Come ha detto il Ministro: è stato approvato in Commissione il nostro - riferendolo a se stesso - provvedimento di legge.

purtroppo così non è stato: abbiamo visto, in effetti, che la capacità del Governo per questioni politiche di accogliere emendamenti, pur essendo in prima lettura, è pari a zero. ho detto prima, l'ordine del giorno approvato, in questo caso - come ho chiesto prima a fronte dell'emendamento 8.0.205 aveva l'unico obiettivo, Vice Ministro, di impedire un aggravio di burocrazia a chi le regole già rispetta.

Vede, vice ministro Olivero, e lo dico anche al suo collega del Ministero della giustizia, si fanno continuamente leggi in questo Paese pensando che così si possano soddisfare le esigenze di repressione del crimine. Scriviamo tante cose, e forse anche troppe, mentre ne basterebbe una. Settimo comandamento: «non rubare». Inizia e finisce tutto lì. Il resto sono declinazioni che semplicemente rischiano, come spesso avviene,

il giudizio su come il Governo avrà recepito anche questi stimoli.

sia con il Governo che con la relatrice, e per questo già precedentemente avevo annunciato il voto favorevole del Gruppo AL-A, che ribadisco ancora oggi.

bersagliare le aziende a partita IVA, o comunque coloro che lavorano serenamente e tranquillamente e pagano regolarmente

Per combatterlo, insieme a una doverosa iniziativa repressiva, occorre favorire la piena modernizzazione di quegli ambiti che non riescono a fare filiera, costruire consorzi e valorizzare la qualità del prodotto, facendo leva solo sul contenimento del costo del lavoro. ci hanno ampiamente ricordato, dobbiamo lavorare soprattutto per rimuovere le cause che favoriscono la presenza dei caporali. Occorre mettere in campo meccanismi trasparenti e di garanzia per imprenditori e lavoratori per far incontrare domanda e offerta di manodopera. Occorre dare al settore quei servizi - dai trasporti, agli alloggi - su cui i caporali costruiscono la loro indispensabilità. Allo stesso tempo, dobbiamo stare attenti a non penalizzare le aziende sane e oneste con inutili o addirittura dannosi aggravi burocratici o - peggio ancora - ritenere che l'intermediazione tra domanda e offerta sia considerata a ogni costo una forma di sfruttamento di caporalato. La prima versione del provvedimento era davvero troppo rigida e si correva il reale pericolo che un'interpretazione restrittiva portasse a definire caporalato ciò che non lo è affatto. Se a questo si aggiungono gli aspetti penali e le pene severe introdotte con il disegno di legge in esame, il rischio era davvero quello di dar vita a processi lunghissimi e a contenziosi costosi e interminabili che, soprattutto nel caso della piccola proprietà contadina, avrebbero scoraggiato molti a impugnare i provvedimenti ingiusti o esagerati. Sempre da questo punto di vista, rimane un'eccessiva rigidità sull'iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Su questo punto, io, il senatore Berger e altri colleghi abbiamo presentato uno specifico emendamento,

che, pur salvaguardando la validità dell'obiettivo, intendevano circoscrivere nella giusta cornice il reato di sfruttamento e manodopera, evitando di affrontare un problema complesso con l'emotività.

per noi sono fonte di perplessità su un provvedimento che nasce sotto le più nobili intenzioni per un problema che va assolutamente contrastato, ma che in alcun modo deve introdurre un clima punitivo e di sospetto verso le aziende sane, che sono la stragrande maggioranza. Prendo atto con soddisfazione che sono stati accolti sia in Commissione che in Assemblea alcuni nostri emendamenti, per la verità simili a quelli presentati da altri colleghi, che hanno parzialmente ridotto il rischio insito nella versione originaria del provvedimento. In particolare, sono soddisfatto per aver confermato la periodicità trimestrale del versamento dei contributi agricoli unificati per non costringere gli agricoltori a sostanziose anticipazioni, così come per la proroga al 2018 dell'entrata in vigore del sistema Uniemens e, infine, per la rinuncia all'introduzione di insidiosi indici di congruità. In futuro si lavori sul fronte dei servizi, così come è stato chiesto dalle organizzazioni agricole, che ringrazio per la collaborazione e l'esperienza che ci hanno fornito. Si lavori per regolamentare in maniera efficace l'intermediazione buona tra domanda e offerta di manodopera e per favorire la piena modernizzazione di quegli ambiti, che vivono un ritardo clamoroso rispetto al ruolo e alla funzione che l'agroalimentare nel suo complesso può dare per la ripresa economica.

per semplificare la burocrazia, che, soprattutto per le piccole aziende di montagna, costituisce un vero e proprio ostacolo. Dobbiamo incentivare il ricambio generazionale, valorizzare i marchi di qualità, favorire la multifunzionalità, incentivare la ricerca e tutto quello che va nella direzione di prodotti sempre più salubri e rispettosi dell'ambiente e rendere, infine, le nostre aziende sostenibili dal punto di vista economico. Con questo auspicio, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento in

Il nuovo articolo 603 del codice penale, che punisce non solo il caporale, ma anche il datore di lavoro, è cosa utile e - secondo me - necessaria, così come l'accoglimento di alcune richieste del sindacato.

Purtroppo, però, dobbiamo anche dire che c'è tanto lavoro da fare e, soprattutto, c'è bisogno di chiarezza. Intanto, per chi non lo sapesse - mi rivolgo al Governo - è notizia di poche settimane fa che l'Italia si è aggiudicata il terzo posto in Europa nella classifica per il per il numero assoluto di schiavi. Inoltre, rispetto ad altri Paesi - è sempre notizia di poche settimane fa - l'operato del Governo è stato giudicato insufficiente nella lotta contro lo sfruttamento.

che svolgono. Noi ci eravamo impegnati tutti a far sì che, se proprio bisognava dare degli incentivi, venissero dati alle agenzie pubbliche. Da questo punto di vista mi sono sforzato

Non vorrei vedere fra qualche mese, dopo i *voucher*, dopo la precarietà selvaggia e dopo i buoni pasto, qualche altra sorpresa, come in tempi passati abbiamo già visto. Lascio un punto interrogativo su questo e, se vogliamo fare una riflessione seria, noi di Sinistra Italiana saremo sempre disponibili da questo punto di vista.

È un provvedimento questo che - senza accusare di retorica l'espressione che sto per usare - riveste davvero una importanza fondamentale per il nostro Paese, che investe l'intera concezione dell'attività primaria, in termini di produttività ma, soprattutto, di compatibilità sociale e di svolgimento del pieno rispetto dei diritti delle persone e dei lavoratori. Io credo che in quest'Aula conosciamo tutti le condizioni davvero molto difficili in cui spesso si svolge il lavoro nei campi;

l'anno scorso almeno quattro braccianti hanno perso la vita nei mesi più caldi e ciò ha provocato - se non altro - un aumento delle ispezioni. delle persone e del caporalato riguarda una platea più ampia rispetto al 2015: le statistiche ci parlano di circa 30.000-50.000 lavoratori interessati in più,

Alla base di questo fenomeno di sfruttamento vi è una distorsione della filiera produttiva: la sfida senza limiti sui prezzi fa sì che siano schiacciati coloro che sono in fondo alla catena produttiva. È un circolo drammatico che può essere rallentato e arrestato responsabilizzando tutta la filiera sull'importanza della qualità nel ciclo produttivo e cercando di agire sulle aziende meno responsabili e di ottenere il sostegno e l'appoggio delle aziende più responsabili, e il cammino che in Commissione abbiamo svolto va esattamente in questa direzione. Io vorrei dare atto al lavoro che in Commissione agricoltura è stato fatto da parte di tutte le forze politiche. Desidero ringraziare ancora una volta la relatrice per la sensibilità dimostrata,

di numerose associazioni e rappresentanze di forze sindacali e aziendali, come anche del mondo dei consumatori e dell'opinione pubblica. Signor Presidente, colleghi, quello in discussione non è il primo intervento legislativo che viene realizzato. Già il Parlamento e il Governo sono intervenuti più volte nel corso di questi anni, a partire dal 2011, quando fu inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro. Nel 2014, e quindi nel corso di questa legislatura, è stata creata la rete del lavoro agricolo di qualità e nel 2015 è stato approvato il disegno di legge oggi in discussione, che ha introdotto strumenti operativi a livello amministrativo e penale. Il 27 maggio di quest'anno è stato anche firmato un protocollo d'intesa che prevede una iniziativa sperimentale di assistenza ai lavoratori nei territori del Sud d'Italia. quindi a dire che è un fenomeno da tempo all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento, ma che ha reso necessario il nostro intervento. Qualcuno ha sottolineato la fretta con cui avremmo agito. Non credo che si possa accusare di fretta il lavoro che abbiamo svolto. Certo, era nell'ottica del nostro intervento la volontà di arrivare a una approvazione dell'Assemblea prima della stagione estiva,

indicano la necessità di un intervento che sentivamo doveroso e che oggi vogliamo varare con un voto che mi auguro più ampio delle forze di maggioranza all'interno di quest'Aula, per dare un messaggio forte a tutti gli operatori d'Italia. Abbiamo fatto, credo, un buono lavoro: variamo un provvedimento che costituirà un segnale molto forte, in attesa

come ogni estate, a memoria d'uomo, la ferita del caporalato si fa più profonda, perché sale in superficie il terribile retroscena di un'economia sommersa, che si serve della povertà per infliggere violenze sistematiche e vessazioni, in una spirale che assume i connotati di una piaga che sanguina, che è la schiavitù che deriva dal caporalato. La sottrazione dei documenti, le condizioni igienico‑sanitarie estreme, gli accampamenti di fortuna e la totale assenza dei più elementari servizi sono solo le evidenti premesse di un doloroso fenomeno endemico, radicato e, per assurdo, connaturato alle nostre campagne, alle coltivazioni, alle colture. A questo, poi, si aggiungono il degrado urbano, l'abbandono umano e materiale e il pericoloso rischio di diffusione di focolai epidemici; condizioni che più volte abbiamo avuto modo di vedere di persona, non ultimo lo scorso 10 luglio a Nardò, in Puglia, in Provincia di Lecce, in un'area che davvero è riduttivo definire un ghetto. Ma ce ne sono tante altre e in tutta Italia, perché questo non è un fenomeno solo del Sud. Ma andiamo per ordine. Questo in esame è un testo che, fin dall'inizio, ha mostrato delle fragilità, a partire da una stesura delle disposizioni che è cambiata fortunatamente - sotto diversi aspetti e rispetto al testo iniziale nel corso del tempo, ma che abbiamo voluto correggere fin da subito con un'attività emendativa incalzante. Devo dire che, sebbene questo provvedimento sia stato presentato il 28 gennaio di quest'anno, sei mesi fa, la maggioranza ha preferito ridursi all'ultimo per capire cosa fare e come muoversi, salvo poi recepire e assorbire alcune o gran parte delle istanze di modifica del Movimento 5 Stelle, anche spacciandole per proprie sotto forma di emendamenti della

Ci tengo a precisare, tuttavia, che questo è solo un piccolo passo in avanti per il mondo del lavoro e dell'agricoltura e ovviamente ci auguriamo che non rimanga l'ultimo, ma sia l'inizio di un percorso che possa andare anche molto oltre, che possa definire quanto viene comunque preso in considerazione riguardo al fenomeno del caporalato. Sì, perché contrastare il caporalato, come fa questa proposta del Governo, è importante. Noi, tuttavia, ci teniamo a significare le nostre proposte, cosa avremmo voluto effettivamente, come avremmo strutturato un disegno di legge. Prima di tutto, le norme del codice penale in materia di caporalato si possono scrivere in altri centomila modi o in diverse formulazioni. Ma, se non cambiamo i fattori reali, quelle norme rimarranno solo formule vuote, senza significato. In un sistema in cui si contano 430.000 lavoratori irregolari solo per il comparto agricolo, l'efficacia deterrente di una norma severa può essere un punto di partenza, ma - come dicevo prima - non certo quello di arrivo. Si doveva poi dare centralità ai lavoratori, restituendo loro - e solo a loro - la dignità che il caporale prima e il caporalato dopo gli hanno tolto, giorno dopo giorno. Inoltre, sin da subito abbiamo richiesto specifiche agevolazioni all'interno delle misure dei piani di sviluppo rurale e sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza lavoro; contenuti che il Governo, sebbene ci sia stato un intento di adesione della relatrice in tal senso, ha voluto un po' laconicamente accogliere in termini di impegno a valutare la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura. Abbiamo sempre detto che occorrono appositi interventi normativi per favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali riguardo ai servizi di trasporto per i lavoratori agricoli che devono raggiungere i luoghi ove prestano la loro attività. E su questo pende un preciso dovere assunto dall'Esecutivo, che non potrà schivare facendo finta di niente. Sempre riguardo al trasporto, abbiamo chiesto l'adozione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti le modalità del trasferimento, e in particolare: l'obbligo per i trasportatori - ovviamente non devono aver subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - di stipulare un'apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

Per noi è necessario attivare un numero telefonico nazionale anticaporalato, che permetta di denunciare i fenomeni di sfruttamento e maltrattamento durante lo svolgimento del lavoro o la conduzione dell'azienda; il tutto in pieno anonimato e prevenendo ogni possibile atto ritorsivo nei confronti del bracciante. Sul piano strettamente tecnico, inoltre, sin dalle prime battute abbiamo contestato con forza la formulazione iniziale della confisca per equivalente, perché due sono le cose: o la norma è stata scritta male o il Governo si era accidentalmente dimenticato di riprodurre l'inciso «anche indirettamente o per interposta persona», oppure c'è stato un inspiegabile tentativo di depotenziare lo strumento della confisca con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ci saremmo trovati infatti davanti all'assurda situazione in cui al condannato sarebbe stata irrogata la pena detentiva pecuniaria prevista, ma non gli sarebbero stati poi sottratti i soldi fatti alle spalle dei lavoratori sfruttati, se fosse stato così furbo da affidarli a un altro. È un vero e proprio obbrobrio normativo che - per fortuna - abbiamo scongiurato, grazie anche alla relatrice che ha accolto pienamente le nostre proposte, facendole proprie. perciò la pena ripetere con forza che le cose che servono o che sono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, devono essere sempre confiscate, salvo, ovviamente, che appartengano a persone estranee al reato. Quando questo non sia possibile, è fondamentale che venga disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato, senza se e senza ma. grande attenzione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che, purtroppo, ad oggi, ha come unici interlocutori le imprese e non i lavoratori. La Rete dovrebbe diventare sinonimo di qualità in modo da poter indirizzare in maniera deterrente, e nello stesso tempo efficace, le verifiche ispettive. Le imprese virtuose, perciò, quelle che - tanto per fare un esempio - applicheranno ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali, dovranno essere invogliate ad aderire, attraverso palesi benefici in termini di incentivi, detrazioni e sgravi contributivi, come quello di un euro per ogni giornata lavorata.

È opportuna l'istituzione di un apposito marchio di qualità per prodotti della Rete, oltre che campagne informative per incentivare l'acquisto di tali prodotti. Ci sono poi la cabina di regia e le cooperative agricole, ma sono i braccianti braccianti che devono poter beneficiare di un'assistenza sanitaria, in modo che lavorare nella raccolta dei prodotti agricoli non debba per forza essere sinonimo di morte. In Puglia, in Calabria, in Campania, come in tutte le terre dove le agromafie si infiltrano, spesso l'unico salvagente a disposizione dei braccianti sono le associazioni. Ma non è possibile affidare a loro e solo a loro

avere una fissa dimora e possano eventualmente puntare sul riconoscimento della loro dimora. Mi avvio alla conclusione, citando solo pochi dati: una montagna di soldi sporchi, che oscilla tra i 14 e i 17 miliardi di euro l'anno e che, per la sola agricoltura si aggira tra i 2 e i 5 miliardi 5 miliardi di euro. Questo è quello che può pregiudicare il caporalato; è importante però non perdere di vista nessun obiettivo. Detto questo, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul testo in esame, ma, ancora una volta, noi riteniamo che questo sia solo il primo passo di una lunga serie, di una lunga maratona. Questa lunga maratona dovrà portare ad un traguardo che possa salvaguardare tutte le persone che fanno parte di questo esercito degli invisibili, perché bisogna assolutamente considerare che queste persone contribuiscono a portare avanti l'eccellenza e la salvaguardia del *made in Italy*. Quindi il Movimento 5 Stelle

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'ordine del giorno reca disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Quello dell'intermediazione illecita e del lavoro sfruttato è un tema piuttosto serio, che ha risvolti talvolta drammatici, ma che tuttavia rimane sotto silenzio. Si tratta del cosiddetto fenomeno del caporalato, diffuso tra le campagne del nostro territorio, Il caporalato rappresenta una forma illegale di reclutamento e di organizzazione della manodopera, specialmente agricola,

e somme illegali, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collegamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali. Pagamento a cottimo, assenza di un regolare contratto di lavoro, dieci o dodici ore di lavoro giornaliero, per un bacino di lavoratori di circa 400.000 persone. Sulla base di queste considerazioni, il Governo ha ritenuto necessario intervenire, attraverso la presentazione di un disegno di legge di propria iniziativa, che risale al gennaio di quest'anno. Ci troviamo oggi a votare in prima lettura su un provvedimento che ha recepito alcune modifiche apportate in sede di Commissione agricoltura, ma che tuttavia nulla risolve per arginare il fenomeno. La stagione di raccolta è più che avviata.

In più, leggendo le disposizioni che si vogliono introdurre con questo disegno di legge, si delinea un regime fortemente repressivo, peraltro dal profilo incerto; talvolta l'aspetto repressivo non assume i connotati di qualcosa che possa risolvere il problema. di legge introduce modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale che, appunto, tratta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La pena prevista per chi recluta, ma anche per chi direttamente utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è la reclusione da uno a sei anni con multa da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato o impiegato. In teoria, una disposizione del genere sembrerebbe essere in linea con l'obiettivo perseguito, ma se solo si ricorre ad un piccolo esempio ci si rende conto di quanto sia azzardata e pericolosa questa disposizione. Ammettiamo che un tale, sia esso reclutatore o imprenditore, sia giudicato colpevole per aver sfruttato il lavoro di dieci braccianti e che il giudice gli infligga la pena più alta prevista: ciò si traduce in sei anni per ogni lavoratore, ovvero in sessant'anni di reclusione. È dunque opportuno, vi chiedo, che il Senato stia vagliando una legge in grado di configurare una situazione di tale genere? In più è scritto che costituisce indice di sfruttamento, tra le altre, anche la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Nulla di più paradossale. Sotto certi aspetti non siamo d'accordo che si consideri come condizione di sfruttamento, e perciò inquadrabile come fattispecie di reato, una violazione di norme di lieve entità sulla sicurezza e sull'igiene sui luoghi di lavoro anche perché manca una specifica su quali tra queste norme rilevino ai fini del novellato articolo 603-*bis*. Chi ci assicura che una violazione non grave di una norma in materia di sicurezza o igiene non verrà interpretata come condizione di sfruttamento? E questo riguarda Forza Italia che, con alcuni emendamenti, si è impegnata affinché venisse previsto come reato non già lo sfruttamento occasionale o quello derivante, appunto, da norme *minoris generis* ma lo sfruttamento grave e reiterato. Dovrebbe essere preminente, ai fini della rilevazione della rilevazione del reato di caporalato, accertare l'intenzione da parte di chi commette l'illecito, di sfruttare il lavoro altrui, sottoponendo i lavoratori a condizioni miserevoli. Invero, dal tenore della disciplina tracciata da questo disegno di legge, vi è il rischio che venga penalizzato l'intero settore agricolo e che ci sia una caccia alle streghe con conseguenti confische, interdizioni, controllo giudiziario dell'azienda e reclusioni sproporzionate perché frutto di un'interpretazione. Ancora una volta ci troviamo di fronte un Governo che rintraccia il problema, in questo caso il caporalato, ma che non ha le capacità di dare una soluzione effettiva, né tantomeno la maggioranza di quest'Aula si affida al buon senso dei Gruppi parlamentari che propongono alcune modifiche in grado di correggere le storture di un disegno di legge così concepito e che sono state respinte totalmente in Commissione. Neanche un minimo di presa in considerazione e di discussione degli emendamenti per un provvedimento che doveva essere importante, fondamentale e che avrebbe dovuto recepire le istanze di tutti i Gruppi parlamentari. È un fenomeno che sicuramente richiede l'intervento del legislatore affinché ponga rimedio alle situazioni più evidenti ma non certo condividiamo lo spirito, così repressivo, sotteso ad un provvedimento destinato comunque ad essere teorico. Dico «comunque» perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, lo citava prima anche il presidente Formigoni, non è nuovo il tentativo di

Ancora una volta, ho una percezione motivata. Potremmo confrontarci tra un anno, o tra due, e fare un bilancio di cosa ha prodotto questa legge. Ho l'impressione che ci sia più una corsa, ora diventata una rincorsa, più che a risolvere il problema a far prevalere un altro concetto che è quello di dire: ho fatto una legge che risolve il problema, che è tutt'altra cosa. tutt'altra cosa. Oggi come oggi, in quelle situazioni, in quelle regioni, in quelle realtà dove il fenomeno delle mafie ha praticamente sotto controllo

che soffrono solo perché hanno bisogno di un tozzo di pane. Pensiamo anche a cosa fa questo Governo per un'agricoltura che oggi è allo stremo, che sta morendo, per le aziende agricole che oggi lavorano, producono sotto costo,

colleghi senatori, oggi chiudiamo la prima tappa di un percorso parlamentare per l'approvazione del disegno di legge per il contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura, che ha coinvolto, in misura diversa, tutti noi non solo nel ruolo di parlamentari, ma anche le nostre coscienze, come quelle di chi sta all'esterno (imprese, lavoratori e, più complessivamente, l'intera opinione pubblica). Il testo che stiamo per approvare è il risultato di un lavoro complesso, a cui hanno contribuito in tanti: *in primis* il Governo, con la presentazione del disegno di legge, cui è stato annesso il testo proposto dal senatore Stefano; i ministri Martina, Orlando e Poletti e i rispettivi Ministeri che, con determinazione, competenza e sforzo di innovazione, hanno affiancato questo percorso; le Commissioni agricoltura, giustizia e lavoro, che si sono impegnate in modo coordinato e minuzioso; la relatrice che ha guidato l'*iter* con equilibrio e competenza. Credo però che vada detto che il collante che ha consentito di rendere fruttifero il lavoro di ognuno è stata la volontà politica dei Gruppi parlamentari pur nei naturali distinguo, hanno accompagnato con senso di responsabilità e flessibilità il lavoro nel corso di questi mesi e hanno contribuito a costruire tutte le condizioni per giungere al testo finale, che risulta estremamente equilibrato e con elevati contenuti di innovazione in cui tanti di noi alla fine si riconoscono. Ci auguriamo che, con la stessa fermezza e volontà politica, venga agevolato il passaggio successivo alla Camera. L'intermediazione illecita di manodopera reclutata e utilizzata in condizioni di sfruttamento da parte di chi approfitta dello stato di bisogno delle persone, siano esse italiane o straniere, donne, uomini e anche bambini, è un fenomeno complesso e multiforme. Nel nostro Paese è distribuito da Nord a Sud. Viene impiegato in produzioni dal valore aggiunto molto diversificato, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura. Si manifesta in dimensioni molto diversificate e, anche se sulle stime esistono valutazioni diverse, ciò che è certo è che il fenomeno è presente e conosciuto. Il quadro che ne esce è estremamente variegato e abbraccia una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare, per il quale il *jobs act* ha da poco ridefinito le sanzioni (che sono solo di tipo amministrativo e rimarranno in quell'alveo), fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani, da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo comunque a condizioni di di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi, che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo, in condizioni di gravissimo sfruttamento nelle quali la degenerazione può arrivare all'uso della minaccia e della violenza. Se qualcuno aveva qualche dubbio sulla necessità di intervenire in modo organico, con tutti i mezzi (non solo repressivi e d'indagine e controllo, ma anche di prevenzione e di formazione) penso che, nel corso di questi mesi, abbia potuto fugarli. Come è indubbio che non partiamo dall'anno zero sia negli strumenti sia nella lotta. Già nel 2011 veniva inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita, nel più volte citato, anche in quest'Aula, articolo 603-*bis*. Alcune Regioni hanno poi sperimentato progetti per costruire sistemi legali alternativi al reclutamento illegale.

il protocollo di recente sottoscritto con cinque Regioni del Sud e il terzo settore per avviare sperimentazioni nella gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, nell'assistenza sanitaria, nell'inclusione e nella formazione. È di questi giorni poi la pubblicazione del bando del Ministero del lavoro, in collaborazione con quello dell'agricoltura, che stanzia 45 milioni per finanziare piccole e medie imprese che vogliono migliorare le condizioni di salute e di sicurezza. Netta è quindi la volontà politica e istituzionale di affrontare i nodi del problema agendo su vari fronti. Non siamo all'anno zero, ma soprattutto siamo nelle condizioni di avere una visione sistemica del fenomeno e di valutare l'efficacia degli strumenti disponibili per togliere dalle campagne quelle situazioni che nessuno di noi vuol più vedere. Il disegno di legge n. 2217 va in questa direzione. Siamo partiti proprio dalle cause dell'inefficienza dell'articolo 603-*bis* per superare quelle rigidità che lo hanno, di fatto, in questi anni, reso inutilizzato, modulando la fattispecie di reato come pure gli indici di sfruttamento per colpire le varie forme in cui il caporalato si manifesta e riconoscendo che nel lavoro nero e nello sfruttamento in agricoltura è colpevole parimenti sia chi recluta che chi utilizza, anche in assenza di violenza. Si riconosce quindi, per la prima volta, in modo esplicito, la responsabilità dell'impresa che utilizza lavoro nero prevedendo attenuanti per chi «si adopera per evitare che l'attività delittuosa delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori». Vogliamo creare delle falle profonde all'interno del criminoso sistema, vogliamo destrutturarlo partendo dalle radici. La fermezza della nostra volontà sarà già di per sé un un importante deterrente. Il dibattito in Commissione, come pure molti interventi in Aula, è stato ricco e credo abbia consentito ad ognuno ad ognuno di essere più consapevoli di come buon lavoro e buona impresa stanno insieme. Sì, perché in Italia ci sono centinaia di migliaia di aziende agricole, che sono generalmente quelle che danno il maggior contributo all'occupazione e alla produzione di ricchezza, che offrono lavoro regolare e adeguatamente retribuito, che si sono innovate, spesso mettendo in comune fasi della lavorazione e della commercializzazione, ed hanno superato i limiti che la piccola e piccolissima dimensione pongono alla competitività. Queste sono le imprese del *made in Italy* di cui dobbiamo continuare ad occuparci. Questa è la sfida che vogliamo affrontare anche con questo provvedimento. Esiste un'agricoltura che aggrega l'offerta, che investe in innovazione tecnologica, che usa la meccanizzazione come sinonimo di sicurezza del lavoro e di salute. Molte delle mansioni in cui oggi vengono impiegati i lavoratori sfruttati, in molte aree dei Paese sono già state sostituite da macchine. Un esempio significativo è la raccolta del pomodoro: nel distretto del Nord non esiste più la raccolta a mano e le imprese stesse hanno costruito quella filiera che mette insieme al lavoro buono la buono la redditività del settore primario. È questa la strada giusta per contrastare in modo definitivo il caporalato nel nostro Paese: sostenere la modernizzazione del comparto agricolo significa non solo superare le arretratezze dei sistemi produttivi, ma anche migliorare il mondo del lavoro. Ciò vale però anche per il sistema pubblico che, oltre a mettere a disposizione strumenti repressivi dei comportamenti delittuosi e a rafforzare e a rendere più selettivi i controlli, deve facilitare l'accesso delle imprese alla legalità, riappropriandosi di quegli spazi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento della manodopera hanno trovato terreno fertile per l'assenza di un'offerta legale e sostenibile di servizi. La rivisitazione della Rete del lavoro agricolo di qualità va a coprire questi spazi. Molti mi hanno chiesto: perché partire dall'agricoltura per affrontare un provvedimento contro lo sfruttamento del lavoro nero? Molti, anzi, si aspettavano un atteggiamento di difesa da parte del settore, ma non è stato così. Il settore sta affrontando la sfida facendosi promotore di iniziative propositive. L'agricoltura si è messa alla testa di questa sfida e oggi siamo qui ad approvare a larga maggioranza questo provvedimento, che segna che segna anche un cambio di passo nei rapporti con la politica e le istituzioni. Questo deve vederci ancora più impegnati nel continuare a sostenere quel percorso di rinnovamento già avanzato, cominciando a condividere, anche tra di noi, un linguaggio che sia più idoneo a un comparto così dignitoso e combattivo.

un ringraziamento davvero sentito, da parte del Governo tutto, alla relatrice, senatrice Gatti, per il grande lavoro profuso durante l'esame del provvedimento.

La relatrice, senatrice Zanoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

Il decreto-legge al nostro esame si inserisce ormai nella buona consuetudine di discutere i provvedimenti in materia di enti locali durante il mese di luglio con l'obiettivo di fornire un quadro di maggiori certezze per gli enti locali, in particolare per la predisposizione dei bilanci per l'anno successivo. Il provvedimento contiene un insieme articolato di misure che interessano tra l'altro le modalità degli enti territoriali concorse al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure principali novità per tipologia di ente. Per le Regioni sono stati previsti 74 milioni in più per il trasporto pubblico locale; è prevista l'assegnazione alle Regioni virtuose delle risorse rinvenienti dalle sanzioni versate dalle Regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio; si da attuazione ai recenti accordi tra Stato e Regione siciliana (attribuzione di risorse Per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane, che sono oggettivamente un livello istituzionale che in questo momento sta soffrendo, per questa fase di transizione prolungata, è prevista la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2015. Si prevedono 48 milioni di euro per il funzionamento delle funzioni fondamentali delle Province e 100 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Si stabilisce la ripartizione della riduzione di spesa corrente tra Province e Città metropolitane e, infine, si limita l'obbligo del pareggio di bilancio 2016 alla sola sede del rendiconto. tratta di misure indispensabili, affinché tali enti possano sopravvivere. Per i Comuni si prevedono una nuova modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con una logica di tipo perequativo, l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità per il 2015 e si stanziano 80 milioni di euro in quattro anni per i Comuni colpiti da sentenze esecutive. inoltre definiti gli aiuti agli enti locali in crisi finanziaria e si prevede la continuità di aiuto ai Comuni calamitati di Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania e Toscana.

infine il piano triennale di stabilizzazione dei maestri nelle scuole materne e negli asili nido, di cui si è tanto parlato, anche in questi giorni, sui giornali. Le misure del decreto-legge in esame fanno seguito, come accennato, ad un complesso di interventi rivolti agli enti territoriali, come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità per il 2016. Nel loro insieme, tali misure hanno come obiettivo il superamento della situazione straordinaria apertasi durante il periodo di maggiore crisi economica e di finanza pubblica del nostro Paese, che ha visto gli enti territoriali dare un fondamentale contributo al risanamento e il ripristino delle normali condizioni di programmazione della propria attività. Dal 2015 è iniziata una nuova politica nei confronti degli enti territoriali, incentrata su un più efficace dialogo istituzionale con gli organismi di rappresentanza, sulla diminuzione dei tagli lineari, su maggiori spazi finanziari di manovra, in particolare dal lato delle spese per investimenti, e su regole di bilancio meno stringenti che in passato. In questo quadro complessivamente positivo, in evoluzione e miglioramento, emergono però ancora esigenze che non potevano trovare spazio in questo decreto-legge, ma che il lavoro della Commissione ha voluto sottolineare, in particolare con l'approvazione di un ordine del giorno della relatrice approvato all'unanimità. Per quanto riguarda i Comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale, che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme, che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione ora che si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane si è da più parti evidenziata la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa,

Si tratta di portare a termine un insieme di interventi in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge n. 56 del 2015. Durante l'esame del provvedimento in Commissione, numerose proposte emendative hanno evidenziato possibili soluzioni a gran parte delle problematiche che ancora riguardano gli enti locali, con un ordine del giorno concordato, riassuntivo delle varie posizioni, il Governo si è impegnato a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti; e anche su un ripensamento e un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale che, forse, a sette anni dalla sua parziale applicazione, forse richiederebbe un ripensamento rispetto anche al tipo di norme che sono state emanate in questi anni. Alle misure per gli enti territoriali in questo provvedimento si aggiungono altre misure. In particolare, su sanità e farmaci vi è un complesso di disposizioni innovative che ridisciplinano alcuni aspetti della spesa sanitaria e farmaceutica. Sul'ambiente: dà la possibilità dell'utilizzo delle risorse per la bonifica delle discariche abusive e si affronta il tema della depurazione delle acque urbane reflue. In agricoltura, sono stati stanziati dieci milioni per sostenere i produttori di latte e dieci milioni per il fondo derrate alimentari per persone indigenti, è previsto un contributo per le aziende suinicole e tre milioni per il fondo per le imprese cerealicole. Tra le altre misure vi sono quelle per il disastro ferroviario di Andria: 10 milioni per i familiari delle vittime e i feriti gravi. Vi sono norme per la predisposizione di strutture di accoglienza temporanea per i minori stranieri non accompagnati. Ancora, sui vigili del fuoco: 193 assunzioni; 400 posti in più in dotazione organica; dieci milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dispositivi di sicurezza per i vigili. Si tratta inoltre di un provvedimento molto atteso dai cittadini e dalle imprese che hanno debiti tributari: è previsto un nuovo piano di rateizzazione. Sulle fondazioni lirico-sinfoniche sono state previste misure di sostegno e revisione degli assetti organizzativi e di ripianamento. Infine, un tema molto discusso sui giornali in questi giorni che viene affrontato È stata data una proroga delle concessioni in attesa del riordino complessivo della materia, per ottemperare anche a una richiesta dell'Unione europea. Consegno agli atti la relazione completa che passa in rassegna in modo più preciso tutti i provvedimenti e passo subito alle conclusioni. conclusioni. Il decreto-legge si inserisce nel più ampio quadro delle innovazioni sia strutturali sia congiunturali che riguardano gli enti locali in questi ultimi anni e che stanno progressivamente delineando un percorso di normalizzazione dell'attività. La conoscenza delle regole e la certezza delle risorse a disposizione consente agli enti locali di programmare la propria attività e di rispettare le regole stesse. E per noi è fondamentale, perché gli enti locali sono la nostra possibilità di arrivare a tutti i territori del nostro Stato. Si tratta di un lento ritorno alla normalità procedurale, anche se resta da affrontare con coraggio in particolare la situazione dei bilanci di Province e Città metropolitane. Concludo con i ringraziamenti, che non sono solo di rito, ai componenti della Commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, per la volontà a discutere nel merito il provvedimento. Ringrazio gli uffici della Commissione e l'ufficio legislativo del mio Gruppo per il solito indispensabile apporto tecnico. Ringrazio il Governo, che, stante l'impossibilità di approvare approvare emendamenti, ha preso impegni con maggioranza e minoranza per l'accoglimento di diversi ordini del giorno in materia di enti territoriali e per il contributo fornito alla ricerca delle soluzioni. Infine, mi rivolgo a tutti i senatori perché valutino positivamente il provvedimento nel merito, fortemente atteso dagli enti destinatari e dai cittadini. *(Applausi

il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione richiede comunque che «l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate che richiedono interventi oggettivamente eterogenei». Esaminando il provvedimento in discussione, per l'ennesima volta notiamo come in un decreto-legge

sanzioni economiche per Province e le Città metropolitane che non hanno rispettato il Patto di stabilità, di discariche abusive, dello Statuto della Regione siciliana, di interventi per gli enti locali in crisi finanziaria per il personale insegnante ed educativo,

Quella era una situazione d'urgenza alla quale, tra l'altro, non è stata data quasi nessuna risposta. Capisco che vi possano essere situazioni di urgenza riguardanti le calamità naturali.

quasi a voler raffazzonare un po' di provvedimenti alla fine del mese di luglio e nei primi giorni di agosto e a cercare di far passare provvedimenti nei quali, magari, mettere dentro un po' di tutto;

Ma, signori, la decretazione d'urgenza è un rimedio previsto dalla nostra Costituzione; già i Padri costituenti pensavano potesse crearsi una problematica nella gestione di uno Stato.

Signor Presidente, ancora una volta sono costretta - come abbiamo detto in Commissione e ci dispiace - a fare un intervento di rito; un intervento un po' sconfortato, perché non è banale violare sistematicamente la Costituzione, non è qualcosa di cui quest'Assemblea e la nostra Commissione si dovrebbero vantare. La collega Stefani ci ha fatto un primo richiamo d'ordine. Questo provvedimento - e ringrazio la collega Zanoni per averlo così correttamente ed esaustivamente illustrato potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per gli enti territoriali ove avesse una natura strutturale. Ma purtroppo una natura strutturale non ce l'ha. Sappiamo che almeno da cinque anni a questa parte, da quando si è cominciato a celebrare questo matrimonio contro natura tra Patto di stabilità e pareggio di bilancio, che ha fortemente impoverito

queste perdessero parte della loro cifra di assistenza ai cittadini per l'incapacità di combinare i due fattori, ciò di cui veramente si sarebbe avvertita si sarebbe avvertita la necessità sarebbe stato un provvedimento destinato non a strappare mancette e benefici contingenti al limitare del generale agosto, ma a dare una spina dorsale, un architrave, una struttura di assistenza agli enti che, in assoluto, hanno sofferto di più per i tagli di questo Governo. Dalla relazione della collega Zanoni possiamo tutti desumere la natura disomogenea di questo decreto-legge; un provvedimento che va dalle discariche abusive a cui si cerca di mettere qualche pezza a colori, come si dice in alcune Regioni d'Italia - alla giusta, doverosa (ma certamente non prevalente in una valutazione costituzionale del provvedimento) necessità di risarcire i territori colpiti da calamità naturali, anche alla produzione di specifiche merceologiche lattiero‑casearie e cerealicole; alla produzione di beni culturali e artistici. Non c'è bisogno di dire altro, non voglio sottrarre altro tempo a questa Assemblea; non c'è bisogno - se non attraverso i titoli - di dimostrare che questo provvedimento non può tenersi insieme. Come giustamente ricordava il collega Morra in Commissione, non è più eterogeneo, è disomogeneo; è caratterizzato da una dismorfia naturale. Sono provvedimenti che non hanno nulla a che vedere gli uni con gli altri e che si affiancano a un'altrettanto naturale assenza - io la considero profondamente innaturale, anzi contro natura - di quei requisiti di necessità e urgenza

perché rappresenta una temporanea e contingente maggioranza. Questa è una violazione profonda del cuore delle disposizioni costituzionali, che noi continuiamo a perpetrare, quasi che il farlo, il creare giurisprudenza di Commissione e di Assemblea, possa modificare in miniera subliminale il senso della Costituzione. Non è così.

la giurisprudenza costituzionale. Non lo farò di nuovo anch'io, perché ormai se potessimo avere un centesimo di euro per ogni volta che abbiamo citato la giurisprudenza della Corte costituzionale, e lo destinassimo a un fondo a vantaggio della povertà, potremmo fare ricco qualcuno. Sappiamo benissimo che la Corte costituzionale ci dice che non esiste una generica urgenza nel provvedere; che la necessità e l'urgenza devono essere debitamente motivate; che non possono essere utilizzati strumenti governativi per creare per creare disposizioni disomogenee. Colleghi, tutti noi, il legislatore - noi siamo il legislatore - non possiamo continuare ad avallare questo modo di fare leggi sciatto e inefficiente, che mette gli operatori del diritto nelle condizioni di non poterlo utilizzare. Abbiamo una stratificazione di disposizioni che ormai si contraddicono tra di loro; si modificano: ne facciamo una, la cambiamo la volta dopo. Non serve a nulla. Non serve a nulla. Lo ricordava il collega Amidei prima: fare una legge che si dice essere utile non significa che sia utile ai nostri cittadini; significa solo fare inutili proclami e noi non siamo interessati a fare proclami, neanche in questo caso. altro elemento, ormai quasi passato in cavalleria rispetto a questa valutazione di costituzionalità, è l'attitudine a inserire in questi decreti-legge *omnibus*, in questi provvedimenti vagone onnicomprensivo, anche norme che non hanno un'applicazione immediata, ma che sono destinate ad avere efficacia per gli anni a venire. Secondo voi questo è compatibile con la necessità e l'urgenza connaturate a un decreto-legge? È mostruoso che dobbiamo raccontarci fino alla noia tutte queste cose, violando sistematicamente i precetti dell'articolo 77. Tutto questo è profondamente non solo sbagliato, ma anche dannoso, perché crea la sensazione non solo dell'inutilità del nostro organo, ma anche della difficoltà di utilizzare gli strumenti che da qui dovrebbero uscire come

soddisfazione che dovrà essere presto reiterata con provvedimenti di questo tipo? A cosa è servito, colleghi, la scorsa settimana votare tutti insieme appassionatamente le nuove regole di bilancio, quando si fa una piccola, ruffiana finanziaria finanziaria estiva? Ma non ci siamo detti, poco tempo fa, che l'unica vera finanziaria è la legge di stabilità, la legge d'autunno, che definisce i conti, le poste, le allocazioni,

il decreto-legge come uno strumento di attuazione del suo programma di Governo? Per quanto ancora? Vogliamo degli esempi all'interno di questo provvedimento? Ci siamo sentiti raccontare fino alla nausea che le Province sono state abolite. Sorpresa: le Province vivono e lottano insieme a noi e sono finanziate in questo provvedimento per le loro spese indifferibili.

per difficoltà di coperture, che vengono anch'esse allegramente "overpassate" quando riguardano il Governo e gli emendamenti della maggioranza. Ma voi sapete, colleghi, a proposito di emendamenti, che alcuni degli emendamenti di noi delle opposizioni sono stati respinti alla Camera per carenza - non ci crederete - di attinenza al testo? Vorrei capire con quale parametro si considera, sulla base di questa disformia testuale un emendamento più o meno attinente a questo testo, che a mio avviso ricomprende, ad una prima valutazione superficiale, questo mondo e quest'altro? Quindi, pur nella comprensione del doppiopesismo e del doppiomisurismo, che sempre caratterizzano il rapporto tra maggioranza ed opposizioni, cerchiamo di non esagerare, cerchiamo di non tirare troppo la corda, cerchiamo di non fare finta di voler essere collaborativi, quando poi alla fine il Governo se la scrive, se la canta e se la suona secondo convenienza.

l'inserimento pattizio di una modifica dello Statuto siciliano, di cui parleremo ampiamente in dichiarazione di voto, che non può essere modificato con legge ordinaria (altra

Per questo noi speriamo, signor Presidente, di poterlo fermare, in uno slancio di ravvedimento operoso ed attivo, attraverso la decisione di tutti noi di non procedere

io non so se ormai è di rito, come diciamo sempre ogni volta in Commissione affari costituzionali di fronte a questo tipo di decreto-legge, e quindi il problema è nostro, che poniamo ripetutamente le questioni pregiudiziali, o se invece siamo arrivati veramente ad un punto di esagerazione, da parte del Governo, nel ricorso ai decreti-legge. Penso che in particolare questo decreto-legge potrebbe essere pubblicato in un manuale di diritto costituzionale

dello strumento della decretazione d'urgenza, ed è sempre lo stesso copione che si ripete.

non certo disorganica, ma organica e omogenea, e dovrebbe essere ancorata e motivata

non dire che vi è una espropriazione, ormai pressoché totale, da parte degli Esecutivi, e in particolare di questo Governo, del potere legislativo del Parlamento. Abbiamo

inseguisse la legge da circa vent'anni, il Governo ha magnanimamente lasciato la piena potestà legislativa

anche far passare molto tempo e magari anche avere la navetta che di solito si applica soltanto in questo caso), e tutto il resto, cioè il 90 per cento dell'attività del Parlamento, di fatto occupata dalla conversione dei decreti-legge. Questo significa non solo che c'è un *vulnus* ma che ormai ci troviamo di fronte ad un *vulnus* permanente dell'articolo 70 della Costituzione. Abbiamo avuto una manomissione di fatto della Costituzione, del del potere legislativo del Parlamento stesso e quindi, alla fine, anche della sovranità popolare. In particolare, potremmo leggere tutti

Le disposizioni contenute sono le più svariate. andiamo dall'accoglienza dei minori stranieri (inserita alla Camera), al potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, all'addizionale comunale sui diritti di imbarco, all'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco,

di interventi che non hanno un filo conduttore e non sono legati neanche dal carattere di urgenza. Se esaminiamo il testo articolo per articolo, ci rendiamo conto

l'esproprio, che viene fatto in totale violazione della nostra Costituzione, del potere del Parlamento e la totale assenza dei presupposti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 77. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 93,

è sottoposto un decreto-legge di ben 24 articoli, ma risulta abbastanza evidente, per le considerazioni già svolte, la violazione principale che sottoponiamo all'esame di quest'Assemblea con la questione pregiudiziale che abbiamo presentato è quella dell'articolo 77,

Noi invece notiamo in questo provvedimento una dilatazione disorganica e disomogenea

anche io, a titolo meramente esemplificativo, ne cito qualcuno: si passa da norme che riguardano il potenziamento e la funzionalità del Corpo dei vigili del fuoco a norme che riguardano le procedure di autorizzazione per le apparecchiature che consentono la risonanza magnetica, fino al riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche; potremmo continuare con tanti altri esempi. Come sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto, si tratta di argomenti che hanno una loro dignità e una loro importanza, ma che non possono essere inseriti in un decreto-legge come quello di cui ci occupiamo oggi. dicevo, potremmo continuare con altri esempi: non ho sentito finora citare quello relativo alle concessioni demaniali, che è materia scabrosa, forse difficile anche da trattare

ha riproposto semplicemente una proroga, già contenuta in provvedimenti precedenti e sottoposta anche al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza invece dire - e questo sì che sarebbe urgente al pari della proroga - cosa intende fare in futuro. Abbiamo letto dichiarazioni in cui si parla di nuovo di una legge delega, ma ci siamo dimenticati che la delega precedente è stata fatta scadere sia dal Governo Monti che dal Governo Letta, e che il Governo Renzi non si era posto il problema della scadenza di quella delega ed ha atteso supinamente e in modo inerte gli esiti del giudizio davanti alla Corte di giustizia europea. Oggi invece sarebbe interessante dire a tutti i concessionari non tanto che si propone in modo così semplicistico quella proroga al 2020, ma che, utilizzando gli spazi concessi dalla sentenza della Corte di giustizia europea, si possono intravedere quei motivi imperativi di interesse generale che consentono di tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto

considerata l'eterogeneità della materia e l'elemento sintomatico, già rilevato più volte dalla Corte costituzionale, dell'assenza del presupposto della straordinaria necessità e urgenza.

In questo senso ci confortano ancora una volta il dettato e i principi della Corte costituzionale, e segnatamente la sentenza n. 22 del 2012 che lo ha enunciato in modo eloquente. eloquente. Come rilevato anche da chi mi ha preceduto, l'ulteriore violazione che noi sottoponiamo all'esame di quest'Assemblea è quella dell'articolo 70. Si continua a utilizzare la decretazione d'urgenza in modo così abbondante e penetrante che le le due Camere non si occupano di altro e, quando lo fanno, lo fanno in modo quasi complementare per riempire gli spazi vuoti tra l'esame di un decreto-legge e l'altro.

Io direi che programma di Governo è un'espressione fin troppo altisonante ed enfatica. Si tratta semplicemente di decreti *omnibus* che erogano piccole mance a singoli elettori - la *captatio benevolentiae* verso singole persone o piccole categorie - senza neanche un disegno preciso che potremmo far rientrare in un concetto di programma di Governo.

cercato di introdurre una vera e propria delega al Governo che comprime ulteriormente le prerogative del Parlamento. Ciò è stato più volte oggetto di attenzione e le precedenti pronunce in questo senso dimostrano che

Chiedo alla collega, ancorché non presente in Aula, cosa ci sia di nuovo nel sottolineare una pratica che è ormai consuetudine consolidata di un Parlamento che ha

non soltanto caratteristiche di omogeneità, ma anche caratteristiche di necessità e urgenza. È inutile che ci prendiamo in giro.

decreto-legge n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. I 41 articoli di cui consta il provvedimento (ricordo che dovevano essere 25) contengono disposizioni relative al fondo di solidarietà e alla semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali, nonché misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

poi l'applicazione graduale delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale e le disposizioni sul dissesto delle amministrazioni provinciali, perché c'è stato ripetuto che erano state soppresse le Province, ma poi bisogna intervenire sul dissesto delle amministrazioni provinciali. contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila; disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio del 1998 a Sarno. Badate che, tra le altre cose, a distanza di diciotto anni, interveniamo su un'alluvione che,

che, se prese in considerazione da chi di dovere, avrebbero potuto evitare il disastro. Ci sono poi le disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio del 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

questo all'interno di un decreto-legge, che è uno, semplicemente perché tutti voi, per quanto diabolici, sapete che cosa sia la *reductio ad unum*. È una procedura per cui, scrivendo in lingua italiana, si rende linguisticamente omogeneo qualcosa che spazia però nell'universo mondo mondo e va dall'accoglienza dei minori non accompagnati alle Città metropolitane, fino al sistema sanzionatorio per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei documenti contabili degli enti territoriali e via dicendo. Voglio dunque dunque citare la senatrice Bernini, che ha avuto la gentilezza di citare il sottoscritto, quando in Commissione ha ricordato che, piuttosto che di eterogeneità, si sarebbe dovuto ragionare di disomogeneità,

come dei criminali - e dico bene: «criminali» - su qualcosa che dovrebbe essere centrale, decisivo e sacro per la nostra missione. Noi siamo il legislatore e allora - perdindirindina! - le leggi facciamole come Cristo comanda e come la Costituzione

ovvero un decreto-legge finalizzato a soddisfare esigenze che non potevano essere rinviate al mittente con un «No grazie!». Bisognava soddisfare queste richieste e questo si è fatto.

si potrebbe eccepire un difetto di costituzionalità, per l'ennesima volta. Per questo, senatrice De Petris, c'è una ritualità in tutto questo dibattito, perché questo

non soltanto inonda le Camere continuamente di decreti-legge, per cui noi siamo qui, senza orario di chiusura perché appunto bisogna approvare decreti che altrimenti non potrebbero essere convertiti, a questo Parlamento viola in particolar modo l'articolo 70 della Costituzione, che forse voi non avete intenzione di modificare con 439 parole, esattamente come vorrebbe il nuovo disposto, ma con poche parole: «La formazione della legge è garantita in seconda battuta dal Parlamento, ma *in primis* dall'Esecutivo, che si appropria della funzione legislativa e impone ai Presidenti delle due Camere e anche al Presidente della Repubblica di dimenticare cosa sia la Costituzione». Mi dispiace infatti dire che, se noi avessimo un Presidente della Repubblica fedele e coerente servitore dello spirito della nostra Costituzione, dovrebbe avere anche un minimo di coraggio, rimandando

dal punto di vista dell'urgenza, di molti di essi, hanno parlato i colleghi che mi hanno proceduto nel presentare le loro questioni pregiudiziali. Soprattutto la senatrice Bernini è stata assolutamente puntuale e precisa nell'indicare

ormai l'eccezione di costituzionalità e diventata quasi un esercizio accademico, perché nessuno (per la verità, debbo dire che in passato non era così) prende veramente con attenzione la questione della costituzionalità e la esamina alla luce della Costituzione. favorevole alla questione pregiudiziale QP2, presentata dal Gruppo di Forza Italia, vorrei soffermarmi in particolare sull'articolo 11, che riguarda la Regione siciliana che riguarda la Regione siciliana e che, dal punto di vista costituzionale, la riguarda in maniera eclatante. Noi tutti sappiamo bene che lo Statuto della Regione siciliana è parte integrante della Costituzione e che per modificarne i contenuti occorre una norma costituzionale. Orbene, lo Statuto della Regione siciliana tassativamente indica alcuni passaggi che qui sono completamente violati. Il primo passaggio è quello della percentuale delle imposte dirette che deve essere riconosciuta annualmente alla Regione siciliana:

autodenunciata dallo stesso Governo, e quindi dallo stesso decreto-legge, riguardo a questo aspetto dello Statuto della Regione siciliana. votato della Regione siciliana dice, e la Costituzione riconosce tale principio nel recepirlo, che esso non può essere modificato neanche a seguito di accordi pattizi tra il Governo e la Regione. Addirittura, su questo piano la Regione, la stessa Costituzione e lo stesso Statuto avevano previsto (ed è in carica, ma a questo punto soltanto formalmente) l'istituzione di una commissione paritetica tra Stato e Regione, che dovrebbe esaminare tutte le questioni delle norme di attuazione della stesso Statuto, ma non certo le modifiche statutarie. Dicevo quindi che è assolutamente vietata la modifica delle norme statutarie a seguito di accordo pattizio tra il Governo nazionale e quello regionale.

in parte già positivamente risolti per la Regione in parte ancora da deliberare, potrebbero cubare - come si suol dire - circa 7-8 miliardi di euro. Vi è quindi una svendita chiara e precisa dei diritti della Regione, non solo in termini normativi e costituzionali, ma anche sostanziali. Mi sono permesso di dire - e lo ribadisco senza tema di essere smentito - che in altre circostanze, se si dovesse se si dovesse paragonare questo accordo a un accordo tra privati, qualcuno potrebbe trasmettere le carte a chi di competenza per un'azione di circonvenzione di incapace. Questo purtroppo è avvenuto e i siciliani ne pagano le conseguenze. ancora più evidente, la norma in parola stabilisce non solo che la Regione si prenda questi 500 milioni e rinunci tramite questo accordo a tutti i contenziosi esistenti, ma addirittura indica alla stessa Regione,

il governo regionale, quindi anche l'Assemblea regionale che poi deve decidere sul bilancio della stessa Regione. stabilisce che il bilancio della Regione, a seguito di quest'intervento normativo, debba portare un avanzo di 227 milioni; in realtà,

Dinanzi a questa aggressione da parte dello Stato italiano nei confronti della Regione siciliana, come se non esistesse anche in Costituzione il principio della leale collaborazione tra enti, proprio come se l'Italia dovesse imporre, come forse si faceva ai faceva ai tempi del Medioevo, un trattato non federativo, ma di protettorato contro un pagamento di tributi o contro un versamento di somme straordinarie,

il silenzio assoluto di un'Assemblea regionale che è prona, pur di poter utilizzare qualche euro, al *Diktat* di rinunciare ai contenziosi costituzionali. Una volta si poteva dire, con il riferimento biblico, che si era svenduta per un piatto di lenticchie, ma ora forse non ci sono neanche le lenticchie nel piatto per cui si è svenduta. Il quadro è veramente

Conoscendo anche l'attenzione con cui molti colleghi qui seguono le sorti delle loro Regioni, immagino, se ciò fosse stato fatto nei confronti di una qualsiasi altra Regione, quale levata di scudi, ad esempio dall'Emilia-Romagna o dalla Toscana, sarebbe venuta contro

che sono stati anche Presidenti di Regione e sanno bene che un *Diktat* di questo tipo non si sarebbe potuto fare nei confronti di una Regione a statuto ordinario. XVII)*. Purtroppo piangiamo l'assoluta subordinazione delle classi politiche regionali alle volontà delle segretarie nazionali; piangiamo in questo caso

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016,

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. I Capigruppo hanno stabilito che entro questa sera si concluda la discussione sulla fiducia, per la quale è stata ripartita un'ora e cinquantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo domani mattina a partire dalle ore 9,30. Seguirà la chiama. Al termine del voto di fiducia si passerà all'esame del disegno di legge sugli sprechi alimentari. Il decreto-legge sul processo telematico sarà discusso dall'Assemblea non appena concluso dalla Commissione. Le Commissioni permanenti sono autorizzate a convocarsi durante i lavori dell'Aula per l'esame dei provvedimenti in calendario.

come questo comportamento rappresenti ormai non più un'eccezione, ma una costante di quest'Assemblea parlamentare.

Da poche settimane si è introdotto un altro

l'ennesima prova di una conduzione dei lavori assolutamente approssimativa, senza una strategia e volta solo a tamponare continuamente le emergenze create da questo Governo.

Partiamo dal concetto di Patto di stabilità. Il provvedimento introduce tutta una serie di deroghe e sanatorie nei confronti degli enti locali

poi mettere delle pezze, ma solo una volta che si è sforato il Patto di stabilità, con un evidente atteggiamento scorretto nei confronti degli amministratori pubblici. infatti, a premiare coloro che, per proprie negligenze o per l'impossibilità di farlo, non sono riusciti a rispettare le regole stabilite dallo Stato, dal Governo e dall'ordinamento della contabilità pubblica.

dell'alluvione avvenuta a Sarno, in Campania, nel 1998 con uno stanziamento di 7,5 milioni nel 2016 e altrettanti negli anni successivi, che equivale a 100.000 euro per ognuna delle vittime di questa triste vicenda. E poi c'è un altro provvedimento, che riguarda un'altra brutta vicenda che ha colpito il nostro Paese molto recentemente, ovvero

non c'è nulla? Ciò dimostra una evidente approssimazione nel gestire le calamità da parte del Governo, che non riesce a fissare regole certe e uguali per tutti, per quanto riguarda

assolutamente intollerabile. Anche negli ultimi anni è avvenuta una serie di calamità che ha colpito i nostri territori e ha fatto vittime, calamità di fronte alle quali c'è stata l'assoluta assenza di questo Governo.

in parte possono essere controllati attraverso un'azione di prevenzione finanziata dal Governo. È da troppo tempo che gli stanziamenti non vengono garantiti ai territori, ma anzi si effettuano tagli, in particolare alle Regioni, che non sono più in grado di governare il proprio territorio.

Province e Regioni che ha creato difficoltà di fronte alle quali voi approvate questo testo con una serie di deroghe e di nuove risorse per tamponare le falle. Questo modo di amministrare e di governare le risorse pubbliche è assolutamente inaccettabile. Il Governo opera tagli agli enti locali, e ai servizi essenziali ai cittadini e non promuove una riduzione della spesa dell'apparato statale. È un atteggiamento di comodo del Presidente del Consiglio che si fa bello con i tagli di cui si devono rendere responsabili gli amministratori locali e che spende, spesso anche impropriamente, le risorse messe a disposizione dei cittadini con una tassazione che ha raggiunto ormai livelli insostenibili. Per tutti questi motivi e per molti altri, signora Presidente, la Lega Nord conferma il proprio voto di sfiducia al Governo, che ormai da troppo tempo non rappresenta più la maggioranza degli italiani e che verrà messo alla prova, finalmente, con un voto vero del popolo nei prossimi mesi, in autunno, con una occasione straordinaria per dire no

provvedimento, che riguarda la mia Regione di provenienza. La scorsa settimana con il mio collega Fabrizio Bocchino abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'accordo truffa siglato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio, che equivale a una vera e propria appropriazione indebita in danno delle casse della Regione siciliana; un accordo che fa acqua da tutte le parti, come ammesso dallo stesso assessore al bilancio della Regione siciliana, che priva la Sicilia di circa sette miliardi di euro, e parliamo di una regione povera. L'accordo contiene ben due violazioni dello Statuto siciliano - come il collega D'Alì ha prima puntualmente segnalato - che limitano gli introiti fiscali derivanti da IVA e IRPEF per un valore di circa sette miliardi, cifra indicata dallo stesso assessore in una intervista a «L'Espresso» in cui, con una certa sfacciataggine, ha ammesso tutta l'inconsistenza dell'accordo. In tutto questo la Sicilia è sull'orlo del *default*. L'economia stenta a ripartire, la disoccupazione è ai massimi storici: un'isola in ginocchio che il Governo guarda solo per costruirci i termovalorizzatori probabilmente per pagare debiti a parti sociali ben definite - mortificando ulteriormente la naturale, ancorché disattesa, vocazione turistica di questa terra, che rimane ancora il fanalino di coda di tutto il Paese. Lo Stato, come qualsiasi usuraio, toglie alla Sicilia i fondi che le spettano per Statuto, per restituire solo una parte, di fatto, purché rinunci alla sua autonomia. tutto questo è stato realizzato in casa PD, impegnando le istituzioni, servendosi in modo distorto delle norme, e per legare le stesse istituzioni. Nessun parere è stato richiesto agli organi della Regione. Non è stata interrogata la Giunta. Non si sono espressi l'Assemblea e neanche gli uffici. Il presidente Crocetta è andato da solo: un sedicente Presidente della Regione siciliana, uomo solo, ostaggio di un partito che non lo ama, ma che lo mantiene per timore di elezioni e dal quale, per il modo in cui ha governato, non ha nulla da sperare. La parte più tragica è che l'accordo prevede che quest'elemosina di 500 milioni (i soldi siciliani concessi da Renzi alla Sicilia) dovrà essere restituita con gli interessi, operando nuovi tagli già previsti nei disastrati bilanci regionali. Attenzione: disastrati dal Partito Democratico,

L'Italia sta facendo alla Sicilia lo stesso servizio che l'Europa ha fatto alla Grecia - ti do i soldi necessari per chiudere i bilanci, al prezzo di un commissariamento di fatto con una sola differenza però: in Grecia il *waterboarding* lo ha fatto la *troika* ad Alexis Tsipras, un uomo coraggioso, difensore del suo popolo; in Sicilia il Governo del Partito Democratico lo fa ad un suo esponente, difensore di sé stesso.

Questo Governo ha ispirazioni antiparlamentari e autoritarie neanche tanto velate. La stessa controriforma costituzionale, che il ministro Boschi va propagandando come panacea di tutti i mali, dal terrorismo internazionale al mal di schiena, è un modo non per cambiare verso come a Renzi piace dire - ma per rendere irreversibile un cambiamento già avvenuto con il crollo democratico dei partiti e leggi elettorali come il Porcellum e l'Italicum che ne è figlio: un Parlamento sfogatoio e capro espiatorio, su cui far ricadere l'incapacità di risolvere i problemi concreti dei Governi e di quest'ultimo in particolare. Signora Presidente, io userò i pochi minuti a mia disposizione per richiamare l'attenzione

perché con un emendamento, e quindi con una modifica presentata alla Camera, si introduce di fatto una delega al Governo in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. non tenendo conto, tra l'altro, del fatto che questa delega al Governo era già contenuta nell'articolo 34 del disegno di legge in materia di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che è stato stralciato in Commissione, chiaramente su richiesta dei partiti di maggioranza, poiché il Ministro aveva assicurato che, stralciando tale articolo, avremmo poi avuto presto un provvedimento *ad hoc*.

c'è bisogno di provvedere. Io mi chiedo come mai dall'inizio dell'anno, quando abbiamo ascoltato il commissario straordinario Pinelli, che è venuto a riferirci la sua ultima relazione semestrale, il Governo si svegli a luglio 2016 e si renda conto di tutta questa emergenza, fino al punto di spingere un parlamentare della maggioranza alla Camera dei deputati a presentare un emendamento che riordina la materia, e quindi contro ogni logica parlamentare?

quello che potrebbe succedere al 31 dicembre 2018, e cioè che le fondazioni lirico-sinfoniche siano alternativamente distinte in fondazioni lirico-sinfoniche e in teatri lirico-sinfonici. Quindi, di fatto, potremo assistere alla suddivisione di queste istituzioni in enti di serie A e di serie B, perché poco ci è dato sapere dei requisiti che potranno avere le fondazioni e quelli che avranno, poi, i teatri lirici e sinfonici.

ai danni del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, senza distinguere chiaramente a chi dette misure saranno destinate. Nel testo dell'emendamento, infatti, leggiamo «al personale anche direttivo» e, quindi, possiamo presupporre che queste misure punitive potranno colpire anche il contingente di personale che non ha di fatto alcuna responsabilità nella gestione delle fondazioni. Allora noi ci chiediamo: ma perché? Cosa ha fatto il personale che non è coinvolto nella gestione diretta delle fondazioni per meritare eventualmente misure punitive? E poi ci chiediamo: ma siamo ancora alle misure punitive? Perché, invece, non prevediamo misure atte a promuovere iniziative e comportamenti virtuosi all'interno delle gestioni delle fondazioni lirico-sinfoniche? Ciò che è, infatti, mancato in tutti questi anni sono le gestioni virtuose, che nulla hanno a che vedere con i componenti delle orchestre o con il personale che lavora all'interno delle fondazioni e che - ribadisco - non ha alcuna responsabilità nella gestione delle fondazioni.

3*-sexies* ha l'ambizione di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione, con decreto ministeriale, dei criteri e delle modalità di erogazione dei fondi per lo spettacolo dal vivo, i cosiddetti fondi fondi appartenenti al fondo unico per lo spettacolo. A seguito di questo decreto-legge, nel luglio 2014 è stato emanato un decreto ministeriale, che ha creato non poco scompiglio nel mondo dello spettacolo dal vivo, per una criticabile e opinabile operazione di introduzione e di utilizzo di un algoritmo che ha fatto sì che molte realtà culturali del nostro Paese, qualificate, accreditate e di riconosciuto merito, si siano ritrovate, dall'oggi al domani, a non vedersi erogati i contributi. Si tratta di realtà culturali che promuovono la cultura sul tutto il tutto il territorio nazionale, a tappeto, in modo capillare e diffuso e questo è importante per contrastare il degrado sociale del Paese. Il

a ottobre con un Consiglio di Stato che non è più in grado di emettere alcun parere, poiché già superato da quanto contenuto in questo comma. E aggiungo ancora che il comma 3*-sexies* ha

nessuno dei due presupposti: né ambiguità di interpretazione, né controversia giurisdizionale, ovvero non ci sono sentenze che si contrappongono. Infine, la norma andrebbe in violazione del diritto di difesa, ex articolo 24 della Costituzione, perché interviene a giudizio in corso e, quindi, cambia le carte in tavola, quando c'è un Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sulla sospensione di una sentenza del TAR. Questo modo di procedere è inaccettabile per due motivi: anzitutto siamo di fronte all'ennesimo sgarbo istituzionale, ovvero non si tiene conto di quello che si fa in Parlamento, e soprattutto si rischia di violare la Corte costituzionale e un articolo della Costituzione. Ditemi voi se questo è modo di procedere. colleghi, siamo in presenza oggi dell'ennesimo decreto-legge giunto dal Governo, e non possiamo non sottolineare che il sistematico ricorso a decreti-leggi e fiducie, fiducie e decreti-legge, e decreti-legge, svilisce il ruolo del Parlamento e, quindi, della rappresentanza popolare. Ciò che appare evidente fin da subito, leggendo il testo, è l'enormità di argomenti inseriti: una sorta una sorta di decreto *omnibus* in cui si parla dei più disparati argomenti che vanno dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco alla rateizzazione dei debiti verso Equitalia, dallo stanziamento di finanziamenti per le imprese agricole cerealicole, ai contributi per la prima casa per coloro che hanno visto distrutte le proprie abitazioni in seguito al terremoto del 2009 a L'Aquila. In particolare, in questo specifico decreto-legge, facciamo fatica ad accettare che argomenti anche molto delicati e importanti possano essere mischiati e trattati allo stesso modo e nello stesso tempo con altri di ben minore rilievo. E tutto questo avviene senza alcuna approfondita discussione di merito né nelle Commissioni competenti né in questa Assemblea, visti i tempi ristrettissimi. Il provvedimento affronta argomenti, tematiche e situazioni completamente diverse tra loro, tutte mescolate in una sorta di calderone e senza alcuna connessione reciproca. Pur di mettere una toppa qua e là, il decreto-legge produce il risultato di soluzioni del tutto improvvisate ed estemporanee a una enormità di problemi, evidenziando, quindi, un modo di procedere abbastanza superficiale e carente di una precisa strategia. Questo non è un modo efficace - a nostro modo di vedere - di affrontare le questioni, tanto è vero che rimangono tuttora irrisolti i problemi che continuano a bloccare il Paese, fra i quali una tassazione eccessiva, una burocrazia asfissiante e una economia, purtroppo, ancora troppo debole. Veniamo al dettaglio di qualche punto contenuto in questo provvedimento. Assistiamo nuovamente alla riapertura della rateizzazione dei debiti verso Equitalia. Si perpetua così la vessazione nei confronti dei cittadini italiani, dato che coloro i quali non pagheranno due rate, anche non consecutive, su 72 rate totali perderanno del tutto il beneficio di rateizzazione del pagamento del debito. In un periodo di crisi, nel quale ancora oggi viviamo, permettetemi di giudicare questa misura del tutto irrazionale e inutilmente feroce. La questione è molto seria e richiedeva, quindi, una maggiore con un disegno di legge *ad hoc* che potesse affrontare definitivamente il problema, anziché cercare di mettere una toppa sul buco all'ultimo momento. Altro argomento che viene trattato sono le Province e le Città metropolitane. Il provvedimento in questione propone una mitigazione delle sanzioni per lo sforamento del Patto di stabilità. Questo può apparire un fatto positivo, ma, a ben guardare, rappresenta solo un rimedio alle disfunzioni provocate in precedenza dallo stesso Governo con la legge che ha creato le Città metropolitane al posto delle Province, Province, le quali, quindi, continuano a esistere con un altro nome, ma senza che i cittadini possano eleggere direttamente i loro rappresentanti in tali enti. Da senatore pugliese, vorrei soffermarmi anche sulla questione delle concessioni demaniali marittime. Su questo tema non possiamo certo dire che gli ultimi tre Governi abbiano brillato - per così dire - per prontezza di riflessi. Sono anni che si parla di porre mano al riordino complessivo della materia, ma questo termine viene spostato ancora una volta più in là nel tempo. Eppure, è evidente quanto l'Italia, e in particolare le Regioni a vocazione turistica come la mia, la Puglia, abbiano bisogno di chiarezza legislativa in materia, visto che sono migliaia le imprese balneari interessate. A livello comunitario la materia è trattata dalla cosiddetta direttiva Bolkestein, che sancisce il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali a partire dal primo gennaio 2016 e impone di procedere con un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione. Appena due settimane fa, il 14 luglio, la Corte di giustizia europea si è pronunciata stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime siano prorogate in modo automatico, e cioè senza procedure di selezione di altri potenziali candidati in grado di aggiudicarsi tali concessioni. Questa sentenza ci ha spiazzato, ma già a febbraio di quest'anno, quando l'avvocato generale della Corte di giustizia europea si era dichiarato contrario alla proroga indistinta e automatica fino al 2020 delle concessioni balneari in essere in Italia, era apparso chiaro che la situazione non si stesse mettendo bene per l'Italia. Inoltre, non possiamo non notare che altri Paesi per certi versi simili al nostro, come Spagna e Portogallo, che però economicamente e politicamente hanno un peso in Europa inferiore al nostro, sono riusciti a tutelare le loro imprese balneari e quindi il loro turismo meglio di noi, chiedendo e ottenendo dall'Unione europea una deroga alla direttiva Bolkestein. Durante l'esame di questo provvedimento alla Camera è stato inserito un emendamento per arginare momentaneamente gli effetti della sentenza della Corte europea, ma - come dicevo all'inizio - anche qui si agisce in maniera estemporanea, con soluzioni la cui efficacia è di breve durata e che servono solo a rimandare, invece che a risolvere i problemi. Ma poiché il nostro ruolo in questo Parlamento è di opposizione sempre ragionata e propositiva, mai finalizzata a distruggere, ma sempre a costruire, non mi esimerò dal ringraziare il Governo per due misure assunte e votate all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari. Mi riferisco - ahimè - alla sciagura ferroviaria avvenuta il 12 luglio scorso sulla tratta Andria-Corato e al tragico bilancio di morti e feriti che ne è conseguito. A gran voce abbiamo chiesto alle istituzioni di intervenire per non lasciare sole le famiglie sconvolte da questa tragedia. Apprezziamo, quindi, che siano stati stanziati 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime e per i feriti. Ma ci tengo ad aggiungere che tali stanziamenti a favore delle famiglie pugliesi, la cui vita è stata sconvolta dall'incidente, non è pertinente chiamarli "elargizioni", termine che suona come una sorta di regalo, ma sarebbe preferibile chiamarli in altro modo, forse indennizzi, perché la sciagura avvenuta è stata non una calamità naturale, ma la conseguenza di errori e della mancanza di sistemi di sicurezza automatici sulla linea ferroviaria. Vigileremo insieme affinché questi fondi destinati alle famiglie pugliesi vengano erogati in tempi brevissimi, perché troppe volte abbiamo visto, purtroppo,

contenute in questo decreto-legge, che rappresentano un supporto economico irrinunciabile per tanti nostri concittadini che soffrono. Come vedete, quindi, qualche elemento positivo c'è e lo riconosciamo, ma sul provvedimento nel suo complesso permane il nostro giudizio critico, perché questo disegno di legge appare scombussolato, imposto all'Aula del Senato in tutta fretta e con l'ennesima fiducia, senza la necessaria riflessione prima della pausa estiva. I problemi degli italiani si risolvono non così, ma con soluzioni organiche e definitive.

Si tratta di un insieme di norme per nulla attinenti tra di loro, che vanno a incidere nei settori più disparati, dando così un'ulteriore spallata alla tanto auspicata, ma mai attuata, organicità dell'attività legislativa. Si va dai minori stranieri non accompagnati ai contentini per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha invece una cronica emergenza di mezzi e risorse umane, passando per frammentarie misure per il personale insegnante ed educativo della scuola dell'infanzia e degli asili nido, continuando a ignorare le insegnanti delle GAE infanzia. E, con la scusa del pareggio di bilancio, si vuole regolare il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche secondo nuovi parametri, che ignorano però le risorse interne e le capacità di autoproduzione degli enti lirici e dei teatri comunali. A questa cattiva abitudine dobbiamo aggiungere la volontà del Governo di blindare in Commissione bilancio il testo proveniente dalla Camera; una decisione che è stata l'anticamera di questa scontata e imprescindibile questione di fiducia per imporre ciò che il Governo vuole, defraudando ancora una volta il Parlamento delle proprie prerogative. Fatta questa dovuta premessa, entrando nel merito del provvedimento, mi preme segnalare che stiamo ancora subendo le conseguenze dell'inserimento dell'articolo 11 nel precedente decreto-legge enti locali dello scorso anno, determinando la marginalizzazione delle piccole e medie imprese

consentito invece per la ricostruzione dell'Emilia. E oggi, con l'articolo 3 di questo testo, si prevede l'assegnazione di un contributo straordinario di 18,5 milioni, di cui 16 milioni al Comune di L'Aquila. Esaminando l'articolato, però, non si comprendono le ragioni di quanto previsto. La modifica apportata all'articolo 67-*quater* stabilisce che, decorso il termine stabilito dal Comune entro il quale i lavori

non mediante i procedimenti ad evidenza pubblica, come invece attualmente è in vigore. Si tratta di una norma che ovviamente è contraria a qualsiasi minimo requisito di trasparenza e che sembrerebbe avere come unica giustificazione la volontà del del Governo di far gestire all'amministrazione comunale i fondi della ricostruzione privata con ampia discrezione e sulla base di calcoli politico-elettoralistici. Non dimentichiamo che il prossimo anno a L'Aquila si voterà

ed è stato totalmente respinto. Così come avete respinto un impegno ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché gli enti locali segnalino le irregolarità degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro trenta giorni dalla loro presentazione, prevedendo la liquidazione degli stessi qualora non ci siano segnalazioni di irregolarità a fronte dell'attestazione degli avvenuti pagamenti di tutte le fatture dei fornitori e dei subappaltatori. Già, ma voi, che comodamente e puntualmente ritirate i 5.000 euro netti di stipendio, più i 9.000 di rimborsi spese che non rendicontate, come potete capire? Tra l'altro i Ministri, che hanno anche un'aggiunta, come possono capire le pesanti difficoltà economiche che fanno vivere con queste norme inserite, con leggerezza all'interno di decreti *omnibus* per i cittadini che invece lavorano, hanno sempre lavorato con professionalità e serietà? Ma al Governo non interessa più tutelare i cittadini. Al Governo basta assicurarsi i favori di alcuni cittadini e, soprattutto, gli interessi che possono tornargli.

economia e tutto il nostro territorio costiero. Mi riferisco al tema delle concessioni demaniali marittime. Per quanto riguarda l'articolo 21-*ter*, che amplia l'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, recependo e facendo proprio un emendamento del relatore approvato all'unanimità in Commissione sanità del Senato, non possiamo che esprimere soddisfazione e tirare un sospiro di sollievo anche se, visto il grande lavoro fatto nella nostra Commissione, avremmo avuto piacere di vedere portato a compimento un *iter* legislativo che era iniziato nella legislazione precedente. Quello che conta però è il risultato. È importante che finalmente sia stata data una risposta seria a a chi ha avuto la disgrazia di nascere con malformazioni terribili come la focomelia o l'emimelia non solo per i nati dal 1958 al 1966, ma anche per tutti coloro che, anche se nati fuori dal periodo previsto, possano dimostrare il nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre in gravidanza e le lesioni o le infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Ora si tratterà di porre la massima attenzione nel definire, con il regolamento previsto al comma 4, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide. Passando all'altra materia sulla quale voglio intervenire, ossia quella contenuta all'articolo 24, comma 3-*septies*, relativo alle concessioni demaniali marittime, non posso che esprimere apprezzamento, insieme ai tanti operatori del settore che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato la proroga al 2020 delle concessioni, erano caduti nel panico. Con questo emendamento, in attesa della revisione e del riordino di tutta la materia per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del

della professionalità acquisita, la rideterminazione dei canoni demaniali, l'abbandono di canoni OMI, l'adeguamento delle aliquote IVA agli *standard* turistici, l'abolizione dell'IMU e l'adeguamento degli studi di settore al sistema catastale. Quanto al periodo transitorio necessario per riordinare la materia e mettere in grado i 600 Comuni costieri di disporre di strumenti adeguati alla nuova gestione degli arenili - penso degli arenili (PUA) - e avere finalmente una seria e completa definizione e composizione del demanio marittimo e delle concessioni in essere e di quelle ulteriormente assegnabili, c'è da augurarsi che sia davvero congruo affinché sia messa davvero la parola «fine» a una questione che si trascina ormai da troppi anni e danneggia economicamente tutto il settore e l'indotto relativo. Con questo articolo si salvano anche più di 300 stabilimenti balneari pertinenziali, le cui concessioni sarebbero decadute a causa dell'impossibilità di pagare gli elevati canoni OMI. Il provvedimento è il primo passo del percorso avviato dal Governo per una revisione organica della normativa che, sappiamo bene, non sarà semplice e richiederà un ulteriore e notevole sforzo da parte del Governo in Europa per far capire la peculiarità del nostro sistema turistico balneare, sistema che corre da Trieste a Ventimiglia con caratteristiche che ne fanno una tipologia La Commissione europea continua a erigere muri e sembra che abbia già manifestato al Sottosegretario agli affari europei pesanti contestazioni al disegno di legge di riforma proposto dal Governo Renzi,

il Presidente del Consiglio ne ha tutte le capacità, dato che ha anche affermato di averne la volontà proprio in occasione di una visita a uno stabilimento balneare della Versilia. Perché, come afferma il sottosegretario Gozi, in un contesto in cui il Portogallo vara una proroga di settantacinque anni è molto difficile convincere i concessionari italiani ad accettare un'apertura del mercato che sembra colpire solo l'Italia. Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo

fatto di numerosi ingredienti, alcuni dei quali chiaramente immangiabili, rendendo il tutto indigeribile, se non mortale. Mi limiterò in questa sede ad alcune battute per dimostrare quanto detto in premessa. Innanzitutto, vorrei sottolineare come sia abitudine ormai del Governo prendere provvedimenti già esaminati nelle Commissioni ed inserirli

Ma andiamo con ordine. L'articolo 3-*bis*, comma 2, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012, consente ai commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai Comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto flessibile. Non si capisce perché si siano dimenticati della prefettura di Mantova (e di Rovigo). Forse perché la Provincia di Mantova non è sede emergenziale? Forse a Mantova l'attività di controllo per contrastare le infiltrazione mafiose non serve? Non sarà che Mantova è esente dalla Questo provvedimento mi ricorda tanto la questione degli aiuti ai Comuni di cui al decreto-legge del 19 giugno 2015, n 78, quando all'articolo 12 avete perimetrato la zona colpita e sono stati dimenticati i Comuni della Provincia di Mantova. Poi in tutti i provvedimenti successivi, dove era possibile sono stati presentati emendamenti per aggiungerli fino a che sono stati approvati nel disegno di legge di stabilità. Quanto lavoro per nulla! Altra chicca - questa è veramente molto bella - è il comma 1 dell'articolo 23 in cui si applica il regolamento europeo n. 559 del 2016, e si stanziano 10 milioni di euro per per ridurre la produzione di latte. L'obiettivo - prosegue la relazione tecnica - è quello di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016. Tenete presente che l'Italia produce il 70 per cento del proprio latte, quindi se si riduce anche la quantità, gli altri potranno esportare con maggior facilità avendolo a un costo minore. La relazione illustrativa indica il periodo di riferimento dal 13 aprile 2016 al 12 ottobre 2016, 2016, in parte già superato quindi si sposterà nel secondo semestre. Ma la cosa interessante che vorrei capire è: come si fa a far smettere una vacca di produrre latte? Le si può dare della prolattina. Però ricordo che quando una vacca deve riprendere la produzione, se nasce un vitello ci vogliono ventotto mesi. Quindi la vacca non può produrre il latte in maniera così alternata. Ma dove vanno a prendere questi 10 milioni?

rispettivamente, per la realizzazione di infrastrutture di *e-commerce* e per lo sviluppo di nuovi prodotti. Quindi, da una parte aiutiamo il settore lattiero-caseario con 10 milioni e dall'altra parte glieli togliamo. Ma non è finita qui, perché il comma 6-*bis*, introdotto in Commissione alla Camera, prevede la concessione di un contributo alle imprese che operano nel settore suinicolo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari. E dove andiamo a prendere questi 10 milioni? Le risorse sono reperite sul Fondo di investimenti per il settore lattiero-caseario, previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Le modalità del contributo saranno poi determinate con decreto adottato ai sensi del comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015. Questo è veramente formidabile, veramente formidabile, come lo è l'articolo 23-*bis*, in cui diamo un contributo di 10 milioni al settore cerealicolo tra il 2016 e il 2017. Ma dove si vanno a prendere questi 10 milioni? Sempre utilizzando fondi destinati anche all'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti. Quindi, è sempre il solito gioco delle tre carte che si vanno a mescolare. Voglio concludere questo ragionamento perché è veramente fantastico il comma 6-*quater,* che cambia la quantità di denaro per le quote latte negli anni 2014-2015.

per un fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario. Quindi, a fronte di 30 milioni di euro per l'Unione europea, il nostro Governo ha chiesto agli allevatori 100 milioni di euro, facendo cioè la cresta.

Oggi, visto che i TAR di Parma e di Brescia vi hanno umiliato in maniera pesante dicendo che non potevate fare queste cose, adottate questo provvedimento (cosa per altro risaputa, tanto è vero che l'avevo detto in quest'Assemblea).

farmaco. Intervengo per chiedere attenzione al rappresentante del Governo su questi temi. L'articolo 21 si pone giustamente un problema serio,

l'assistenza farmaceutica ospedaliera sta forando regolarmente il tetto previsto *ex ante* del 3,5 per cento rispetto al fabbisogno complessivo del Servizio sanitario.

Il comma 1 prevede che questa debba essere fatta in base ai criteri già sanciti un anno fa nell'intesa con le Regioni. Purtroppo non possiamo non ricordare che da troppi anni continuiamo a prorogare o comunque a non vedere attuati i provvedimenti che il Parlamento adotta per favorire un maggior controllo della spesa farmaceutica. Ci auguriamo che questa volta i provvedimenti necessari vengano adottati e che non contengano che non contengano elementi di improvvisazione, perché si tratta di miliardi che riguardano la spesa delle Regioni e la salute dei cittadini. Con riguardo alla lunga serie di commi che cercano di affrontare il tema di come sanare il pregresso dello sforamento della spesa farmaceutica, vorrei segnalare alcuni aspetti.

Una cosa deve però essere chiarita, ovvero che si tratta di uno sforamento che riguarda 3,2 miliardi di euro, che si sono accumulati dal 2013 al 2015. Si tratta quindi di una cifra imponente, rispetto alla quale non possono che essere posti alcuni quesiti.

una volta convertito definitivamente il decreto-legge in esame - una posta che le Regioni possono scrivere in entrata; 1,2 miliardi di euro non sono poca cosa, in periodi di grande restrizione per il Servizio sanitario. Che dal 2013 ad oggi ci siano state queste *defaillance* nel sistema di governo è assolutamente da valutare con grande attenzione e credo che dovremmo anche domandarci, in base al principio della responsabilità, quali conclusioni e quali decisioni debbano essere prese. Per il pregresso si trova dunque una soluzione accelerata, che prevede anche uno sconto rispetto a coloro che devono ripianare tale sforamento. una soluzione che, purtroppo, a quanto ci risulta, è già stata oggetto di bocciatura da parte del TAR del Lazio e che quindi rischia di non essere una soluzione definitiva. Ciò ci preoccupa enormemente, così come - lo sottolineo - il *payback*, cioè lo sforamento a carico della filiera della distribuzione e a carico delle aziende farmaceutiche, che per la prima volta

Concludendo, credo dunque che sul governo della spesa farmaceutica ci debba essere una grande attenzione, affinché non ci siano ulteriori ritardi e improvvisazioni.*(Applausi

dopo che già a metà del mese di luglio abbiamo approvato una legge che ha stabilito le nuove regole ordinamentali per la loro contabilità. Anziché creare un clima di certezza normativa e consentire agli enti che governano il territorio di programmare sul lungo periodo i propri bilanci e i propri interventi a sostegno delle comunità di riferimento, si continua a perpetuare un quadro normativo transitorio. A legislazione vigente le regole sono queste, ma non è detto che durino a lungo. Si mormora di un ulteriore contributo alle finanze pubbliche, che verrà richiesto agli enti del territorio, da inserire nella legge di stabilità per il 2017. Quindi, da qui a breve, cambiando il quadro economico-finanziario, anche le regole subiranno ulteriori modifiche. Il decreto-legge in esame, poi, contiene proprio di tutto, come è ormai abitudine del Governo e come tanti colleghi anche questa sera hanno ricordato nel è ulteriormente gonfiato, strada facendo, di articoli e commi, che entrano in un testo già inizialmente assolutamente eterogeneo. Allora, qualche domanda bisogna porsela immediatamente. È mai possibile che per qualsiasi cosa succeda in Italia ci sia bisogno di un decreto-legge? È credibile che non esista una provvista di risorse, nell'ambito del bilancio dello Stato, per poter intervenire in casi di necessità, senza bisogno di un decreto-legge? È pensabile che si debba intervenire su ogni cosa e, ancora, su fatti accaduti nel lontano 1998? É ammissibile che anche norme di carattere ordinamentale debbano essere cambiate in continuazione? Questo è, a nostro avviso, un modo di procedere completamente sbagliato e costituisce una strada che produce solamente incertezze normative e decisionali. Il decreto-legge in esame, lievitato da 25 a 41 articoli, una serie di commi aggiuntivi, dotati comunque di una propria portata normativa, non semplifica la vita degli enti che si occupano del governo del territorio e non risolve i loro problemi. Per quanto riguarda Comuni, Province e Regioni, il problema principale era e resta quello di essere, di fatto, passati dall'idea di finanza propria dei primi anni Novanta a questa idea di finanza derivata a giorni alterni, che è completamente illogica. Ogni mediazione di denaro ha un costo: quando la mediazione avviene in ambito politico e passa attraverso più livelli decisionali, ai costi iniziali si sommano oneri ulteriori. Seguendo quindi questa ondata di antipolitica, che noi legislatori avremmo dovuto contrastare e non assecondare, è addebitata ogni sorta di nefandezza alla gestione dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Quando, al contrario, chi riesce a mantenere una certa obiettività, non può che riconoscere che gli enti di Governo del territorio hanno fatto il meglio di sé, producendo investimenti, infrastrutture e benessere nel momento in cui hanno avuto risorse proprie a disposizione. Certamente vi sono stati alcuni casi di sperpero assurti all'onore delle cronache, ma gli sprechi veri esistono, e continueranno ad esserci, soprattutto a livello della spesa statale, dove il controllo non è prossimo, dove le somme sono più elevate e dove i margini di distrazione sono maggiori. E certamente la nuova china che si è presa ora non premia i Comuni ben amministrati, ma premia quelli governati male, non gratifica i Comuni virtuosi, ma gratifica quelli spendaccioni. Ma sopratutto non vi è alcuna perequazione tra imposte versate e risorse poi ridistribuite ai territori. Risorse e responsabilità sono alla base di ogni buona regola di finanza locale dei territori laddove, sia in Europa che nel mondo, si registrano efficienza e buona amministrazione. E quindi, oltre ad essere un sistema fiscale ingiusto, non innesca quella sana concorrenza tra il buongoverno dei differenti enti del territorio, che è uno dei richiami per attrarre nuovi residenti o nuovi insediamenti produttivi. La mediazione statale, operata anche sui fondi che riguardano i Governi territoriali è ora completamente iniqua. Lo dimostra il fatto che troppe sono ancora le partite finanziarie aperte, ad esempio, tra lo Stato ed i Comuni. Lo dimostra la necessità, oggi, di finanziare le funzioni fondamentali delle Province,

non abbiano risorse. Non è esatto dire che non le hanno. La verità è che le risorse gli sono state tolte da questo ritorno a un neocentralismo della peggior specie. Esso inizia con i tagli ai bilanci degli enti territoriali, sacrificandoli alle manovre di finanza pubblica, prosegue con un incerto ritorno alla finanza derivata e continuerà qualora venisse approvato il quesito al *referendum* costituzionale. Se vincesse il sì, si avrebbe un ulteriore centralismo, che non lascerebbe spazio alla azione dei neo senatori, rappresentanti dei Comuni e delle Regioni cooptati nel nuovo Senato. Essi non avrebbero alcuna reale possibilità di incidere sulle politiche nazionali, ma nemmeno su quelle dei territori che rappresentano. Un'altro luogo comune di questi giorni è quello, più volte ripetuto, che attraverso le modifiche alla legge di contabilità in attuazione della legge rinforzata, conseguente alle novella costituzionale dell'articolo 81, non saranno più possibili interventi micro settoriali o localistici. A parte il fatto che anche con la legge di contabilità vigente tali interventi non sarebbero dovuto essere possibili. Al contrario, noi tutti abbiamo presente quanto accaduto nelle ultime leggi di stabilità che contenevano numerose norme micro settoriali. Ma poi cosa dovrebbe significare quanto appena affermato: che dovremo assistere ad altri decreti-legge, come quello ora in Aula, infarciti di norme micro settoriali o localistiche di ogni tipo, perché non si possono più mettere nella nuova legge di bilancio? Siamo ovviamente all'assurdo! Inoltre non si può sottacere il lungo elenco di articoli e commi aggiunti al decreto-legge al nostro esame, per i quali è stata presentata una tardiva relazione tecnica, che non riesce a fugare i dubbi sulle coperture finanziarie. mai possibile che il Governo che intende digitalizzare la pubblica amministrazione non riesca ad inviare al Senato una relazione tecnica in un formato elettronico pienamente leggibile, anziché una pessima copia via *telefax*? Concludendo, ci troviamo di fronte a norme *spot*, da cui poi non possono derivare misure risolutive dei problemi affrontati. Questo decreto-legge, andandosi a sommare agli altri 50 precedentemente emanati, ci convince ancora di più della inadeguatezza dell'azione del Governo. Il Paese ha gettato letteralmente via trentatre mesi in cui si sarebbe potuto cercare di agganciare quella timida ripresa che ha caratterizzato l'economia mondiale e di cui l'Italia ha beneficiato solo in minima parte. Al contrario, inseguiamo provvedimenti che, nella forma, nello stile e nei contenuti, ricalcano modelli già visti e rivisti, che non hanno aiutato e non aiuteranno a fare andare avanti il Paese.

tutto ciò che dovrebbe servire per avviare una fase nuova per le finanze degli enti locali, che consegni finalmente ai governi del territorio autonomia, risorse, programmazione e responsabilità. Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa Stefano Ricucci è stato nuovamente arrestato per false fatturazioni in un processo tributario truccato, che stava per costare al contribuente (e quindi a tutti noi) 20 milioni di euro. Voi mi chiederete cosa c'entra. C'entra invece. Ricucci è noto alla storia recente del nostro Paese per diverse frasi celebri, celebri, fra cui l'espressione «furbetti del quartierino». Questa è l'espressione che usò per descrivere sé stesso e gli altri cosiddetti immobiliaristi romani nella triste vicenda BNL-Unipol del 2005. furbetti del quartierino sono quelli che pensano che le regole di una collettività siano un impaccio, che solo i fessi debbano rispettarle. I furbetti sono quelli che fanno sì che illegalità e corruzione in questo Paese siano di un livello tale che lo sviluppo e l'occupazione siano inferiori alle nostre enormi potenzialità. Purtroppo, una norma a favore dei furbetti del quartierino è presente nel disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. Non ce l'ho con il Governo. Sto parlando dell'articolo 13-*bis,* introdotto durante l'esame alla Camera. Questa disposizione introduce norme aggiuntive rispetto a quelle previste nel cosiddetto decreto riscossione del 1973,

se la somma è superiore a 50.000 euro, per avere la dilazione bisogna dimostrare la difficoltà economica. Il comma 1-*bis* dell'articolo 19 prevede che, se si dimostra la persistente difficoltà, si possa ottenere un'ulteriore dilazione di altri sei anni (e fanno dodici).

tutto. Ebbene, colleghi, si fa un gran parlare di tagli alle Province, di *spending review*, di inammissibilità di molte proposte di legge per carenza di copertura finanziaria. Non si trovano i soldi per chiudere i tavoli di crisi in giro per l'Italia e per rinnovare i contratti agli insegnanti e ai pubblici dipendenti. Non si trovano i soldi per i Comuni

Noi dipingiamo Equitalia come un mostro. È possibile che vi siano stati burocratismi e rigidità, ma bisogna stare molto attenti quando si lanciano messaggi negativi di questo tipo, anche perché, per restare al tema delle bollette, le imprese energetiche (ENI, ENEL e le altre) non hanno bisogno della

invece, rinuncia a riscuotere i suoi crediti. Avere leggi che consentono dilazioni di pagamento fino a diciotto anni, significa abolire il sistema della riscossione in questo Paese. Se viene smantellato il sistema della riscossione, crolla tutto il meccanismo di cui all'articolo 53 della Costituzione.

Anzitutto, vi sono imprese che lavorano legalmente e contrattano con la pubblica amministrazione, le quali devono pagare le tasse e, quindi, subiscono la concorrenza sleale di quelle che non pagheranno mai. E poi vi sono le migliaia di lavoratori del settore della riscossione che fanno un mestiere essenziale per la collettività e lo fanno con intelligenza e impegno. Che ne faremo? Vogliamo trascurare i livelli di professionalità e di produttività che essi esprimono e che anche loro diventino un altro comparto di crisi? Insomma, signora Presidente e colleghi, mi auguro proprio che si trovi un rimedio a questo scempio. PRESIDENTE. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta siamo riuniti in quest'Aula per votare la fiducia al Governo. Il conto delle fiducie ormai si è perso e il Parlamento è sempre più privato delle sue funzioni. Sebbene si tratti di uno strumento assolutamente legittimo, un Governo saggio e realmente democratico dovrebbe essere in grado di non abusarne. Ma così non è. Lo sanno tutti. La questione di fiducia, in teoria, servirebbe a combattere l'ostruzionismo. In pratica sta diventando lo strumento in mano al Governo per impedire il dibattito ed evitare il confronto in Aula. Porre la questione di fiducia su un singolo provvedimento significa costringere chi non è d'accordo a votare a favore, contro le sue stesse ragioni. È un punto davvero basso della vita politica e parlamentare di questo Paese, cari colleghi. La fiducia è diventata la regola mentre dovrebbe essere l'eccezione. Vorrei pertanto ricordare al Governo che la Costituzione in vigore non è quella a firma Boschi. È quella dei nostri Padri costituenti, che prevede una doppia lettura dei provvedimenti legislativi. Ad oggi, quindi, la doppia lettura costituisce la regola e deve essere utilizzata per cogliere gli aspetti positivi, quali la ricchezza del dibattito e la individuazione di punti di contatto tra maggioranza e opposizione. Il Governo Renzi, invece, sembra avere un solo faro: la velocità. Ma, come dice un vecchio proverbio, «la gatta frettolosa fa i figli ciechi». Un esempio ne è il nuovo codice degli appalti, approvato tanto velocemente salvo poi dover tornare indietro e adottare dopo appena tre mesi dalla sua approvazione un errata *corrige* che coinvolge 181 articoli su un totale di 220. Ma andiamo all'oggetto della seduta odierna. Il provvedimento oggi in discussione prevede la concessione di una serie di contributi a favore ad esempio - dei territori colpiti dal sisma del 2012 e delle vittime della alluvione del Sarno del 1998. Constato con piacere anche la previsione di spesa di 10 milioni di euro a favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi del disastro ferroviario di Andria-Corato, questione che mi sta particolarmente a cuore, quale *ex* sindaco del mio Comune, Corato in Puglia. Tuttavia, non posso non sottolineare che il provvedimento che stiamo per varare solo in teoria detta disposizioni per gli enti locali. Di fatto, è una sorta di carrozzone in cui è stato inserito ben altro. Direi di tutto. Mi sia consentito un esempio. Con questo decreto-legge si risarciscono i danni legati all'assunzione di un farmaco risalente agli anni Bene, ne sono felice. Ma cosa c'entra con gli enti locali? Questo provvedimento, inoltre, è criticabile sul versante della tempistica. Interviene su questioni attinenti al bilancio degli enti locali, prevedendo modifiche in ordine alla tempistica di presentazione dei documenti di programmazione

Si tratta di disposizioni che accolgo con favore perché tengono conto di quanto la stessa ANCI, nel corso della audizione tenutesi sul decreto-legge in esame, aveva promosso. Ma, allo stesso tempo, sono aspetti che non posso non criticare proprio per la tempistica, come dicevo. Il provvedimento incide su un bilancio non più programmatico ma sul rendiconto, quando ormai i giochi sono stati fatti. sono stati fatti. Se avesse veramente voluto essere di aiuto per gli enti locali, avrebbe dovuto essere adottato non certamente a luglio, ma nel primo trimestre dell'anno. Voglio sottolineare anche altre disposizioni che, nel merito, riducono le risorse a favore dei Comuni, trasformandoli nel *bancomat* del Governo ledendo la loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa, proclamata ormai solo a parole nella Costituzione. Non scordiamoci mai che gli enti locali costituiscono l'istituzione più vicina ai cittadini, quella che più di ogni altra è chiamata a rispondere alle esigenze espresse dal territorio. Ma molto poco si fa per tenere conto di questa sacrosanta realtà e, purtroppo, si continuano a ridurre le risorse a disposizione dei Comuni che, di fatto, sono privati delle necessarie risorse per svolgere in maniera efficace ed efficiente le proprie funzioni. Faccio un altro esempio: con questo provvedimento si attacca il fondo di solidarietà comunale prevedendo che, a decorrere dal 2016, la quota del fondo di solidarietà comunale sia pari al massimo a 80 milioni di euro. Mi permetto di ricordare, cari colleghi, che il fondo di cui stiamo parlando ha la finalità di limitare le disuguaglianze tra i Comuni, ma, se il suo tetto continua a ridursi, è chiaro che l'intento che persegue rimarrà lettera morta. Questo provocherà un danno alle collettività e agli enti locali, che si vedranno ridotti gli introiti a disposizione e saranno sempre più in difficoltà nell'erogare quei servizi che i cittadini richiedono ai Comuni. Mi sia concesso, infine, un ultimo passaggio. Il provvedimento in questione prevede la riduzione delle sanzioni a carico degli enti locali che hanno sforato il Patto di stabilità. Si realizza un assurdo: vengono premiati gli enti locali meno virtuosi, quelli che non hanno rispettato il Patto, a scapito degli enti più virtuosi che hanno osservato tutte le regole.